accaduto questa notte relativo alla nota vicenda legata al ministro Mastella. I deputati de «La Destra», chiedendo a viva voce che il presidente Prodi venisse alle Camere a riferire su quanto accaduto, non ottenendo ascolto hanno occupato l'Aula di Montecitorio. Da quel momento sono stati sequestrati in Aula; sono state chiuse le porte e non è stato consentito loro né di bere un bicchiere d'acqua, né di mangiare un panino, né di recarsi in bagno, con

possono impedire al Papa di parlare in un'università, ma dei deputati, regolarmente eletti dal popolo italiano, non riescono neanche a convocare il Governo per sentire cosa pensi di problemi di nevralgica importanza. Chiedo quindi, proprio per rispetto della dignità dello *status* di parlamentare, che anche lei si faccia carico di stigmatizzare il comportamento dei deputati Questori e del Presidente

Senatore Morselli, per quanto riguarda la presenza del Presidente del Consiglio in relazione alle dimissioni

apre una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Governo sull'emergenza rifiuti in Campania». Ricordo che i tempi del dibattito sono stati ripartiti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e comunicati ai Gruppi. Ricordo inoltre che le proposte di risoluzione o eventuali riformulazioni potranno essere presentate entro un'ora dalla conclusione delle comunicazioni del Ministro.

Governo*. Signor Presidente, premetto che mi soffermerò esclusivamente sulla

sia maturata questa emergenza; la do, in parte, per scontata e ritengo che possa, e debba, essere oggetto di valutazioni da parte del Senato,

Il primo è una crescente difficoltà nell'utilizzo degli unici due polmoni che hanno dato respiro negli ultimi mesi al sistema di smaltimento dei rifiuti in Campania, cioè la discarica regionale di Serre-Macchia Soprana e il sito per lo stoccaggio delle ecoballe di Giugliano-Taverna del Il sito di Macchia Soprana, gestito in maniera inefficiente (e spesso con volontà ostruzionistica), presenta carenze gravi, soprattutto nella stagione invernale. Le soluzioni tecniche apportate hanno consentito di mantenere la discarica aperta ma con un livello di efficienza a fasi alterne. Ciò significa che ogni volta che la capacità di smaltimento di Macchia Soprana si riduce, vi è un corrispondente quantitativo di rifiuti non smaltito.

Il secondo e più grande problema riguarda lo stoccaggio delle cosiddette ecoballe. I cittadini di Giugliano, anche sulla base di un ordine del giorno approvato dal Senato nel giugno scorso, hanno ottenuto dall'allora commissario Pansa la chiusura di Taverna del Re, che rappresentava l'unico sito di stoccaggio provvisorio in funzione in Campania, ove venivano accatastate le ecoballe prodotte dai sei impianti di trattamento della Regione. Sotto la pressione popolare, peraltro gestita dalle Forze dell'ordine senza incidenti di rilievo, si è dovuti arrivare alla chiusura del sito al 31 dicembre 2007. Altro punto alla base del precipitare della crisi è stato il seguente: il commissario Pansa decise, d'accordo con tutti i Presidenti delle Province (che, lo ricordo, erano i subcommissari per l'emergenza rifiuti) di costruire cinque nuove piazzole per lo stoccaggio delle ecoballe sparse nella Regione. Per l'individuazione dei siti fu espressamente richiesta la collaborazione delle Province. Tale collaborazione, come emerge dalla relazione del commissario Pansa del 31 dicembre, non è stata fruttuosa e spesso ha avuto solo un effetto dilatorio. Difatti, nonostante gli appelli del commissario delegato, che richiedeva una mediazione politica con il territorio, le scelte tra novembre e dicembre 2007 sono state compiute quasi tutte dalla struttura commissariale e contestate sia dai sindaci interessati che dalle stesse popolazioni attraverso atti interdittivi e ricorsi giurisdizionali. Le forzature del commissario Pansa hanno consentito l'apertura di un sito di stoccaggio realizzato in provincia di Benevento,

di Lo Uttaro a Caserta sulla base di un provvedimento della magistratura. In tal modo, nell'unica Provincia che si era resa autonoma, si assisteva alla paralisi totale del sistema di smaltimento dei rifiuti. Infine, come sottolineato dall'allora commissario e attuale prefetto di Napoli, Alessandro Pansa, si è diffusa una tendenza, da parte dei soggetti interessati all'emergenza rifiuti, a evitare la cessazione della gestione straordinaria. La relazione commissariale inviata al Presidente del Consiglio il 31 dicembre 2007 evidenzia con chiarezza che man mano che si aveva che si aveva la sensazione che si andava verso l'uscita dalla precarietà si diffondeva una serie di comportamenti tesi a mantenere, invece, lo stato d'emergenza e commissariale. Nella relazione del commissario Pansa si evidenziano interessi convergenti anche di amministrazioni locali che percepiscono la tassa sui rifiuti solidi urbani e non smaltiscono i rifiuti, nonché una serie di interessi assai meno nobili da parte di strutture collegate al ciclo di smaltimento e gestione dei rifiuti stessi. Veniamo agli ultimi interventi svolti dal dal precedente commissario Pansa. Nonostante le difficoltà di contesto, organizzative e operative, il commissario delegato Pansa nei pochi mesi di attività commissariale ha avviato una procedura ristretta accelerata per l'affidamento della gestione del termovalorizzatore di Acerra e dei tre impianti di ex CDR (Caivano, Giugliano in Campania e Tufino) ubicati nella Provincia di Napoli per chiudere il ciclo dei rifiuti; a fine gennaio è prevista l'assegnazione degli appalti. All'inasprirsi della situazione di emergenza nelle scorse settimane, il commissario delegato, in sede di incontri con il Presidente della Regione, della Provincia e con il sindaco di Napoli, ha valutato l'ipotesi di riaprire la vecchia discarica di Pianura al servizio della città di Napoli.

consapevoli degli alti rischi sotto l'aspetto della legalità e dell'ordine pubblico. Per quanto riguarda la legalità, poiché si trattava di una discarica su terreni appartenenti a una società colpita da interdittiva antimafia con molteplici interessi nella zona, sono state adottate tutte le precauzioni possibili d'intesa con le Forze dell'ordine. Per quanto riguarda l'ordine pubblico, a fronte

Passando ora alle azioni del Governo per il definitivo superamento dell'emergenza, a fronte della situazione appena descritta, l'Esecutivo, nella riunione tenutasi a palazzo Chigi l'8 gennaio scorso, al fine di superare in modo definitivo il problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, ha individuato un percorso con obiettivi di breve e medio termine. Va sottolineato che la crisi è concentrata essenzialmente nelle province di Napoli e Caserta, quelle di Benevento, Avellino e Salerno la situazione, pur nella generale criticità regionale, è sotto controllo. Nel breve termine, l'obiettivo è di fronteggiare l'emergenza eliminando, nel più breve tempo possibile, i rifiuti depositati per le strade cittadine. A tal fine si è deciso di nominare un commissario straordinario nella persona del prefetto Gianni De Gennaro, al quale si affianca con responsabilità operative e di logistica il generale di divisione del Genio militare Franco Giannini. Il prefetto De Gennaro, nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio, ha pieni poteri per l'individuazione delle modalità d'intervento e per la selezione dei siti necessari per fronteggiare l'emergenza. Con una nuova ordinanza firmata ieri dal Presidente del Consiglio, il prefetto De Gennaro istituisce un'unità di crisi permanente a Napoli con l'ausilio delle amministrazioni dello Stato coinvolte nella gestione dell'emergenza. Il commissario De Gennaro si avvarrà di personale facente capo alle seguenti aree: area economico- finanziaria, cui è preposto un soggetto attuatore designato dalla Presidenza del Consiglio; area tecnico-operativa, cui è preposto il genio militare del Ministero della difesa; area giuridico-amministrativa, cui è preposto un soggetto attuatore designato dal Ministero dell'interno; area tecnico-impiantistica, cui è preposto un soggetto attuatore designato dalla Presidenza del Consiglio, dipartimento Protezione civile; area tecnico-ambientale e per la raccolta differenziata, cui è preposto un soggetto attuatore designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; area di tutela della salute, cui è preposto un soggetto attuatore designato dal Ministero della salute. La seconda decisione affidata al commissario riguarda l'impegno a definire un nuovo accordo istituzionale con i Comuni campani, le Province e la Regione, così come auspicato dalla Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, che porti a una definizione il più possibile concordata sui siti su cui intervenire. Il commissario ha inoltre il compito di predisporre un piano operativo per assicurare lo smaltimento dei rifiuti, normali e speciali, facendo ricorso sia ai siti immediatamente utilizzabili, tra quelli individuati dalla legge n. 87

il concorso qualificato delle Forze armate per quanto riguarda situazioni di straordinaria necessità e urgenza. Egli deve inoltre definire un piano di sostegno alla Regione Campania da parte delle altre Regioni italiane su base volontaria per queste settimane di emergenza straordinaria. Al momento, attraverso il coordinamento della Conferenza delle Regioni, c'è un'adesione per lo smaltimento di circa 100.000 tonnellate di rifiuti, tra speciale e tal quale, da trasportare gradualmente nei prossimi mesi

Nel medio termine gli obiettivi sono i seguenti: dopo aver ripulito le strade e aperto le discariche temporanee e strutturali (quelle indicate dalla legge n. 87 del 2007), ripristinare la responsabilità del ciclo di smaltimento dei rifiuti agli enti locali uscendo definitivamente dalla logica del commissariamento; dotare la Regione Campania, attraverso procedure straordinarie, di almeno tre termovalorizzatori (Acerra, Santa Maria La Fossa e Salerno). Nell'ordinanza, che ho precedentemente richiamato, firmata ieri dal Presidente del Consiglio, il sindaco di Salerno è nominato commissario delegato per la localizzazione, progettazione e realizzazione dell'impianto di termodistruzione previsto a Salerno, nonché degli impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti e alla raccolta differenziata nel comune di Salerno. Nel medio termine occorre inoltre predisporre le occorrenti misure per la raccolta differenziata dei rifiuti. A tal fine, i Comuni campani dovranno elaborare il relativo piano nei prossimi due mesi; avranno poi a disposizione sessanta giorni per la realizzazione dello stesso piano. La mancata attuazione da parte delle amministrazioni comunali di queste misure nei termini stabiliti, determinerà l'immediato commissariamento dei Comuni inadempienti. Da ultimo, signor Presidente, vorrei ricordare che

e su questo stiamo lavorando in queste ore (sulla falsariga di ciò che avvenne a Milano quando ci fu un'emergenza dello smaltimento), le popolazioni

la fase di brevissimo periodo. Dobbiamo smaltire tutto il pregresso e contemporaneamente produciamo 7.100 tonnellate al giorno di rifiuti. L'avvio di una raccolta differenziata forzata, straordinaria da parte delle popolazioni potrebbe ridurre le 7.100 tonnellate in maniera sensibile e aiutarci ad uscire dall'emergenza.

Segnalo che la qualità della produzione dell'ecoballa campana è giudicata - ahimè dalla magistratura, non da noi - insufficiente rispetto ai limiti posti dalle leggi vigenti. Ci adopereremo e ci stiamo adoperando in queste ore, anche con l'aiuto delle Regioni, per dotare di impianti di emergenza, cioè rafforzare la capacità di selezione degli impianti esistenti, in modo da produrre un trattamento dei rifiuti adeguato alle normative che ci consenta uno smaltimento sul mercato del CDR, alleggerendo sostanzialmente il problema. È ovvio che parliamo di interventi che non possono avvenire nelle prossime giornate, ma debbono aver luogo nelle prossime settimane.

debbano andarsene, ma credo anche che in questo quadro sia fallita la politica di quelle forze di sinistra che hanno sostenuto e sostengono ancora questa amministrazione. Secondo: esprimo piena solidarietà agli abitanti di Pianura e a tutti i cittadini della Campania che hanno subito tanti inganni, patiscono questo scempio e lottano per il diritto alla salute e alla difesa della propria terra. Terzo: non credo che il Governo abbia un vero piano alternativo; mi pare abbia rimesso in campo solo vecchie proposte e che venga usata l'emergenza per imporre quegli inceneritori pericolosi giustamente contestati dalla popolazione. Quarto: è inaccettabile che, invece di sviluppare fino in fondo un dialogo con le popolazioni, siano stati inviati in Campania un supercommissario, per di più nella figura di un superpoliziotto, e l'Esercito. Quinto ed ultimo credo che l'ultimo vero piano di emergenza sia cominciare da subito non solo la raccolta differenziata, ma un piano di riduzione drastica dei rifiuti. Riduzione, riuso, recupero e riciclo sono gli assi su cui invertire la tendenza,

La relazione che ha svolto il Governo ci trova del tutto insoddisfatti: infatti, è particolarmente lacunosa lacunosa e chiede la solidarietà del popolo italiano nei confronti delle popolazioni napoletane e campane, ma non dice che tale solidarietà si deve coniugare necessariamente con le dimissioni dei responsabili di questa sciagura. Bassolino, la sua Giunta e i responsabili politici della Campania devono fare un passo indietro e consentire che il popolo italiano, chiamato a compiere un sacrificio nome della solidarietà, possa al contempo sperare che il domani sia diverso. Non si può certamente pensare che il dramma causato da questi amministratori domani improvvisamente non ci sia più, se saranno sempre gli stessi a gestire la Allora, le procedure d'urgenza, gli sperperi, la collusione con le cosche malavitose: credo che sia necessario, una volta per tutte, risolvere tutto

in relazione, soprattutto, alla situazione gravissima in cui oggi versa l'intera Regione, una Regione in ginocchio, signor Ministro, senza speranza e senza futuro che rispecchia una Nazione con l'immagine distrutta. Ormai da ogni parte vengono segnalate responsabilità ed omissioni di ogni genere. La stessa Corte di giustizia della Comunità europea, su denuncia della stessa Commissione europea, con una sentenza del 26 aprile 2007, nella causa C13505, ha già avviato contro l'Italia la procedura di infrazione. La stessa Commissione nella sua lettera riconosce che il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, affronta la situazione di emergenza prevedendo l'apertura di quattro nuovi siti di discarica. L'avevamo già detto durante l'estate, signor Presidente. Infatti, la Commissione dichiara che le misure in esso previste appaiono insufficienti a risolvere i problemi strutturali dovuti alla mancanza di una adeguata rete di impianti di smaltimento in Campania, come invece richiesto dal combinato disposto degli articoli 4 e 5 della direttiva europea In particolare, secondo la Commissione europea, il decreto-legge n. 61 si limita a stabilire interventi finalizzati alla rimozione degli enormi volumi di rifiuti accumulati senza predisporre l'elaborazione di un piano strutturale volto ad eliminare le cause prime dell'emergenza ed a realizzare un efficace sistema di smaltimento e raccolta dei rifiuti per il territorio campano. Ora, agli inizi di gennaio, per far fronte all'emergenza e dare sostenibilità al ciclo dei rifiuti, il Governo ha platealmente annunciato l'apertura di tre termovalorizzatori, ad Acerra, a Santa Maria La Fossa e a Salerno, e di un numero sufficiente di discariche tale da consentire l'autosufficienza regionale a medio termine nella gestione dei rifiuti, oltre al concorso qualificato delle Forze armate nelle situazioni di straordinaria necessità ed urgenza per il rapido superamento dell'emergenza il cui utilizzo dovrebbe essere oggi attualizzato e concretizzato. Signor Ministro, abbiamo ascoltato attentamente la sua relazione. Il quadro disastroso della Campania è sotto i suoi occhi come sotto quelli di tutto il mondo. Più di un decennio di cattiva gestione e di omissioni gravissime da parte dei vari commissari gridano vendetta. Lei stesso ci ha fornito un quadro desolante della situazione attuale e passata. Il Governo che lei rappresenta non ci ha dato alcuna assicurazione seria per l'immediato futuro. La sua è stata una dichiarazione di resa su tutti i fronti:

Allo stato attuale delle cose non credo si possano suggerire idonee soluzioni. Non ne terreste conto. Ma adesso, signor Ministro, credo sia giunta

Non siete ancora contenti dei disastri che avete combinato? Credo sia veramente giunto il momento, signor Ministro, di andare a casa, di passare la mano. Dovete

è quello di lasciare il passo ad altre forze che veramente potrebbero risolvere la situazione. Voi l'avete incancrenita, seguendo determinati *iter* legislativi di cui poi non avete tenuto conto. Mi riferisco al citato articolo del decreto-legge.

Signor Presidente, signori senatori, questa dovrebbe essere una discussione che riguarda la Campania e i suoi rifiuti. In realtà la Sardegna ha avuto dei "rimbalzi"- così possiamo definirli - di questa tragica situazione veramente negativi. Una bella mattina i sardi si sono svegliati e hanno appreso che una nave era partita da Napoli e trasportava a Cagliari i rifiuti e trasportava a Cagliari i rifiuti campani. Quanti rifiuti? Quali rifiuti? Dove li avrebbero trasportati? Perché questa iniziativa? Nessuna risposta è stata data ai sardi; si è solo saputo che il governatore della Sardegna Soru si era recato a Roma e, per motivi ancora imprescrutabili, aveva consentito questo trasferimento. Lo aveva consentito in violazione della legge regionale sarda 24 aprile 2001, n. 6, che fa divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire nel territorio della Sardegna rifiuti urbani non pericolosi. Questa legge era stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale in un giudizio svoltosi inizialmente di fronte al TAR della Sardegna. con la sua sentenza n. 12 del 26 gennaio 2007 aveva dichiarato che questa legge sarda, che vieta di portare in Sardegna rifiuti urbani non pericolosi, è stata dichiarata legittimamente costituzionale; è una legge che non viola la nostra Costituzione. Ci siamo chiesti e abbiamo ancora insistito per sapere perché il governatore Soru ha adottato quest'iniziativa che vìola una legge. Vorrei aggiungere che la solidarietà è qualcosa di importante,

che la Sardegna non ha mai avuto l'impressione, nei momenti di grande bisogno, che ha attraversato e ancora attraversa, di godere della solidarietà del resto dell'Italia.

sostengono il dovere nazionale di aiutare ad alleviare la grave emergenza campana, ricordando anche che moltissimi rifiuti moltissimi rifiuti industriali provenienti dall'Ipca di Ciriè trovarono, a suo tempo, ospitalità legittima nel territorio campano. Questi cittadini, però, sostengono, aggiungono e ritengono che tutto ciò debba comportare a suo tempo un'esplicita assunzione di responsabilità, anche con atti formali, delle autorità di Governo nazionali, locali e del commissariato fino

l'assunzione anche delle responsabilità personali sia ciò che fa la differenza, che dà credibilità ad una nuova stagione, che ricostruisce un rapporto di fiducia con le popolazioni. È stato pubblicato ieri

e non posso non ricordare quella discussione del maggio dell'anno scorso, con l'ampia audizione di tecnici, personaggi politici, assessori, presidenti e sindaci

dobbiamo essere messi nelle condizioni di sapere cosa votiamo, di essere sicuri dei piani che sono proposti e della fattibilità delle azioni di intervento che sono state suggerite. Noi abbiamo criticato duramente il commissario, ma fortunatamente adesso diamo pieni poteri ad un nuovo commissario. Abbiamo infinitamente sollecitato la cogestione delle Province, abbiamo esaltato un piano regionale, ma la cogestione delle Province, dal mese di maggio ad oggi, non ha prodotto nulla di differente e significativo che abbia sbloccato la situazione.

Ora, se nessun soggetto politico istituzionale è riuscito a risolvere tutto questo, nell'anno in cui il Governo è stato chiamato a decidere e ad assumersi duri impegni politici e finanziari, è del tutto evidente che va accolta la dimensione assolutamente eccezionale

ma di un'attività che è stata fallimentare e che ha portato la Regione Campania nel baratro.

Tutte le comunità che hanno dovuto ospitare i siti hanno giustamente manifestato il loro sdegno ritenendo, e - secondo me - a giusta ragione,

sono convinto che per incanto si risolveranno tutti i problemi. Le Province devono risolvere, ciascuna per la propria

Il superprefetto (così è stato definito), il grande servitore dello Stato (anch'io mi associo a queste affermazioni) non può con la bacchetta magica risolvere problemi atavici e strutturali.

molto elevato nelle persone che vivono in quella zona. È chiaro dunque che il tema del monitoraggio, nel quadro complessivo delle discariche abusive presenti in Campania, della loro bonifica

ha dichiarato che le attuali violazioni della legislazione comunitaria per quanto riguarda la gestione del ciclo integrato dei rifiuti potranno portare quanto prima all'applicazione di sanzioni e di multe al nostro Paese. È già stata avviata una procedura di infrazione nel giugno scorso che andrà avanti. Secondo il Ministro per le politiche europee si tratterebbe eventualmente di una condanna che porterà il nostro Paese a pagare da 20.000 a 70.000 euro al giorno. È una spesa insostenibile, ma soprattutto sarebbe un ulteriore degrado del modo con cui il nostro Paese partecipa allo sforzo comune all'interno dell'Unione Europea per il risanamento ambientale del territorio.

o per comunicazioni del Governo a seguito di ordinanza, come questa volta, in meno di due anni, sempre sullo stesso tema: i rifiuti in Campania. in quattordici anni di emergenza non si può più parlare di straordinarietà: siamo alla normalità. C'è un'assenza totale dei poteri locali che oggettivamente pesa moltissimo nella risoluzione del tutto questo ha generato una sfiducia totale ed una esasperazione enorme nella popolazione. Come non guardare con preoccupazione

discariche illegali su tutto il territorio, che hanno portato a migliaia e migliaia di rifiuti tossici nocivi provenienti dalle Regioni prevalentemente del Nord, del Nord, provocando una situazione di allarme sanitario, tanto che anche gli indici di alcune ASL ci dicono che c'è un'incidenza del 28 per cento in più di tumori in alcune parti del territorio campano rispetto alle altre Regioni d'Italia.

risparmiando sui costi di normale smaltimento e gestione. A ciò si è aggiunto il disastro del ciclo dei rifiuti, inesistente per come è gestito in Campania.

che è sicuramente un provvedimento utile; nello stesso tempo, però, dobbiamo anche rimettere in moto un processo di credibilità delle istituzioni locali, che hanno dimostrato nei loro governi una propria incapacità a risolvere il problema.

Di qui è originata una cessione di sovranità da parte degli enti locali e della Regione agli industriali, agli impiantisti, alla FIBE, a chi ha fatto un appalto unico mettendo nelle mani di un'unica impresa la responsabilità di governare il ciclo dei rifiuti.

che gli stessi enti commissariali sono enti di spesa improduttiva per gli obiettivi da perseguire. Gli stessi commissari che hanno messo in moto il meccanismo dei consorzi obbligatori per la raccolta differenziata, espropriando le amministrazioni comunali, non hanno apportato nessuna soluzione a questo problema, anzi, l'hanno aggravato. Infatti, i consorzi non fanno raccolta differenziata e impediscono ai comuni virtuosi di farla per proprio conto.

o di terremoti. Lo sgombero dei rifiuti dalle strade non sarà possibile se non si realizzerà una solidarietà nazionale da parte delle Regioni e già alcune hanno iniziato un lavoro positivo con il Governo e con la stessa Regione Campania.

che non si decida immediatamente il loro superamento. Relazioni dello stesso Governo riferiscono che siamo in presenza di un autentico malaffare, che lì ci sono davvero gli aspetti del clientelismo che incancreniscono tutta la situazione e, addirittura, che essi agiscono in contrasto con i poteri locali;

La stessa unità di crisi, che giustamente è stata costituita presso la Presidenza del Consiglio, credo sia un ausilio importantissimo al fine di dare un contributo al piano di risanamento e di bonifica, l'altro aspetto indispensabile per rendere chiara la volontà del Governo di tornare alla normalità, ma una normalità che sia garanzia di trasparenza e democrazia per quelle popolazioni.

su quest'intervento ho riflettuto a lungo, perché ero quasi tentata di rileggere quelli che ho svolto in quest'Aula,

che lui soleva sempre affermare che i problemi non possono essere risolti dalla cultura, dalla mentalità che li ha prodotti; ritengo, invece, che noi abbiamo continuato a veder perseverare questa cultura.

assistito ad una situazione veramente incredibile nella città di Napoli e in Campania, devo dire che la maggior parte degli osservatori si è esercitato nell'additare l'ambientalismo e gli ambientalisti come la causa della situazione a cui si è arrivati.

a monte, noi, che vediamo come funziona da altre parti ed anche nelle Regioni più virtuose, ci ritroveremo sempre in una situazione di emergenza.

alla nota gara di cui tanto si discute.

sul banco degli accusati vengono posti coloro che avevano denunciato per tempo quegli imbrogli, anche perché certamente - diciamolo con chiarezza - quella non fu una gara limpida

sul collo e dobbiamo risolvere la questione di chi debba smaltire le ecoballe, perché per l'ultimo anno e mezzo certamente è spettato allo Stato e alla Regione, ma per tutti gli anni precedenti - com'è noto - dovrebbe spettare alla FIBE.

non certamente casuale, per far sì che l'emergenza alimentasse l'emergenza e che non ci fosse pianificazione, per poter continuare a sperperare e gestire situazione in modo straordinario, deresponsabilizzando completamente le amministrazioni locali. prego, concluda,

Onorevoli colleghi, signor Ministro, cercherò di svolgere un intervento pacato, anche se mi riesce difficile dopo il comizio della collega De Petris, che ha richiamato episodi del passato sui quali vi sarà modo di intervenire in altra seduta. Vorrei guardare al futuro e soprattutto svolgere alcune brevi considerazioni, dato il tempo a disposizione, su un concetto, quello

delle altre Regioni e in nome di questa solidarietà è stata chiamata in campo anche la Regione Abruzzo. Signor Presidente, signor Ministro, vorrei anzitutto che ognuno di noi facesse mente locale alla distinzione tra la solidarietà e l'altruismo: non è il caso di fare lezioni in quest'Aula (non ho né i titoli, né la capacità, né il tempo per farlo), ma si è solidali quando si condivide con altri qualcosa di cui si è titolari in misura sufficiente; si è invece altruisti quando, come si vuol dire, ci si toglie il pane di bocca e si dà ad altri quello che invece serve a se stessi. Ebbene, in questo caso le Regioni sono state chiamate ad uno sforzo di altruismo e in particolare la Regione Abruzzo che, voglio ricordarlo, collaborerà nello smaltimento delle 100.000 tonnellate di rifiuti da portare al di fuori della Campania per un ammontare di ben 15.000 tonnellate tonnellate di rifiuti. Il 15 per cento di questa quantità è accollata ad una Regione che ha una popolazione poco superiore al 2 per cento dell'intera popolazione italiana.

se la Regione Abruzzo, come altre, disponesse di discariche o di sistemi di smaltimento dei rifiuti all'avanguardia o comunque più che sufficienti allo smaltimento delle proprie necessità, probabilmente non staremmo nemmeno a discutere; ma in realtà è noto che nel territorio della Regione abruzzese le discariche funzionanti (che sono sole due per due Province sul totale di quattro) hanno un'autosufficienza limitata al 2008. Pertanto, questo carico

sostanze tossiche. Tra l'altro, questo stato di emergenza ormai non si può chiamare più così, perché è diventato una situazione quasi abituale. Si è già verificata un'emergenza alla quale le altre Regioni hanno contribuito e sono state solidali, compresa la Regione Abruzzo; questa emergenza si è ripetuta e temiamo che si ripeta anche in futuro. Vi è quindi un rischio di continuatività dello stato emergenziale, che poi può ulteriormente indebolire il sistema di smaltimento dei rifiuti in tutto il territorio nazionale. C'è poi un argomento di dettaglio che può apparire peloso, ma che tutto sommato ha la sua validità, considerando i tempi magri delle finanze pubbliche, quello del corrispettivo di questa attività di solidarietà, che, per esempio, è rimasto in sospeso per quanto riguarda la Regione Abruzzo e la passata emergenza. Voglio aggiungere soltanto una battuta. Ho apprezzato, nella dichiarazione pacata del ministro Santagata,

dare poi credito ad una Regione come quella abruzzese, che si è pronunciata in consiglio regionale contro la politica dei termovalorizzatori

o anche il Ministro dell'interno, visto che ormai la questione rifiuti ha assunto la caratteristica di emergenza e di sicurezza pubblica.

Nessuna amministrazione è stata mai messa sotto il giogo per il semplice fatto che non sa affrontare un'emergenza. Dalle nostre parti, però, per emergenza si intende un evento imprevedibile, un terremoto, un'alluvione, qualcosa che siamo impreparati ad affrontare; a quel punto scatta anche una grandissima solidarietà locale, regionale, nazionale. Il fatto però che ogni cittadino produca circa un chilo, un chilo e mezzo di rifiuti al giorno e che l'attività principale delle amministrazioni locali sia quella di provvedere all'allontanamento e allo smaltimento di tali rifiuti è tanto ovvio

la responsabilità in via esclusiva dell'insorgenza di un illecito esborso di denaro pubblico alla condotta avventata e negligente tenuta dal commissario delegato

di Governatore della Regione, non poteva amministrare con due tasche in modo alternativo. Le funzioni di commissario erano state assegnate per la risoluzione di un problema, l'emergenza rifiuti, e la gestione della Regione era altra cosa. Non si poteva fare confusione con le due casse.

vorrei brevemente illustrare, non può fare a meno di affermare che siamo di fronte ad un gravissimo problema di igiene e di salute pubblica, nonché di immagine del nostro Paese. Deve essere immediatamente chiusa questa fase commissariale. Quattordici anni hanno comportato grandissimi dispendi e nessuna risoluzione.

primario proprio. Questo perché è molto facile essere buoni, come si è fatto in questi quattordici anni, ma è molto difficile essere giusti. Oggi al Paese dobbiamo dare questa impressione. Dobbiamo dare un senso di giustizia a chi vive in quei posti, che ha diritto a vedere salute e a vivere in modo decente, perché lì non si vive più in modo decoroso. Tutto questo, ripeto, per un senso di giustizia, ma anche di lealtà verso tanti italiani che hanno pagato e sono stati solidali verso la Campania e che poi hanno visto vanificati tutti i loro sacrifici.

non è un'emergenza. È da anni un fatto strutturale che traduce, in modo chiaro e disgraziatamente a tutto il mondo, la disamministrazione che subisce da tempo la regione Campania. Noi parliamo di rifiuti perché sono quelli più visibili, ma c'è anche un'immondizia non visibile. Non mi riferisco soltanto ai rifiuti tossici provenienti da altre Regioni, che per troppi anni sono giunti in Campania dove una magistratura, distratta per le troppe intercettazioni alla Woodcock, non ha disposto i mezzi per far analizzare i suoli delle discariche dove questi venivano venivano accettati, nascosti e occultati. Vi è un'altra immondizia meno visibile, che è il sistema di potere del centrosinistra in Campania. Mi riferisco al sistema sanitario. Oggi è sotto gli occhi di tutti la situazione delle tristi vicende dell'Udeur in Campania e, quindi, della questione della nomina dell'amministratore dell'azienda sanitaria di Caserta e di tutti i fatti ad essa collegati. C'è il problema della sanità in Campania che vede primari e aiuti nominati, di fatto, non dall'assessore regionale alla sanità Montemarano, bensì da un *leader* storico, l'onorevole Ciriaco De Mita. Questa è altra immondizia. È un sistema di potere ignobile che la Campania subisce da tempo. E non dimentichiamo la formazione professionale, una famosa ideologa della CGIL consulente ed assessore alla formazione,

però qui per aver uno scatto di orgoglio è bene che anche la società civile campana si interroghi, perché sono troppi gli esponenti delle organizzazioni sindacali e datoriali, degli ordini professionali e di tanti altri contesti della cosiddetta cosiddetta società civile che, in qualche modo, anziché agire in modo fermo e forte contro la disamministrazione del territorio spesso sono distratti o trovano momenti e convenienze, per le loro attività. Ed allora, per avere uno scatto di orgoglio di questa società campana, ci vuole un elemento scioccante, significativo, peraltro giusto e forse anche tardivo. allora al presidente della Repubblica Napolitano, il quale essendo napoletano non può essere imbrogliato come lo è stato per anni l'ex presidente Ciampi, che recandosi a Villa Rosebery o in pizzeria nel centro storico e trovando le strade opportunamente pulite, dissertava del Rinascimento napoletano anziché preoccuparsi della nostra situazione. Il Presidente della Repubblica conosce bene chi sono questi personaggi che governano il territorio e sa bene che è venuto il momento di dire basta, perché solo così la società civile si potrà ricredere, avere

al Presidente del Consiglio, prima di intervenire in quest'Aula, di non venire con quella faccia da pacione, come ha fatto in televisione, assicurando che le scuole sarebbero state aperte grazie all'Esercito e poi sappiamo che le scuole sono chiuse.

è al 20 per cento, di non prendere più in giro la popolazione. La raccolta differenziata a Salerno è inesistente e, quindi, non c'è un centro-sinistra buono e un centro-sinistra cattivo; c'è un centro-sinistra che deve andare a casa in Campania.

mi domando come mai non sia presente, non dico il Presidente del Consiglio, che ha altri problemi, ma il Ministro dell'ambiente; mi viene il dubbio che voglia tenersi le mani libere per contrastare ancora un'azione commissariale che l'ha visto sempre in prima posizione. Oggi è facile sparare sulla Croce Rossa di questo sistema di potere e sull'incapacità di decidere che ci ha portati a una situazione disastrosa, a una situazione disastrosa, che coinvolge tutto il Paese e ci fa fare delle figure veramente allucinanti a livello internazionale. Voglio ricordare che non più tardi di un anno fa, quando in questa Aula parlavo insieme al mio Gruppo della questione Campania come questione nazionale, le ironie erano tantissime. Forse avevamo visto un po' più avanti già allora; non ne siamo felici, perché, oltre al disastro ambientale che esiste in quella Regione e che è sotto gli occhi di tutti (e qualcuno si ostina ancora a chiamarlo potenziale),

lo dico al Governo e vorrei dirlo anche al Ministro dell'ambiente - che quei Paesi siano più incivili di noi. Forse, visto quello che accade, siamo noi più incivili e forse, con tutto il rispetto, qualche qualche analisi sulla nostra civiltà dovrebbe farla anche il Ministro dell'ambiente, lo stesso Ministro che in Campania é stato eletto. È la sua Regione, vi ha preso i voti, ed in Campania non è riuscito a conseguire nessun risultato, se non quello di enfatizzare una situazione già difficile. Dicevo che è facile ironizzare, ma credo che una politica seria debba passare a valutazioni serie; fare valutazioni serie significa anche trovare soluzioni. già all'atto della nomina del commissario Bertolaso, ha cercato di lavorare per collaborare e per coinvolgere anche la cittadinanza, perché quello che manca è proprio un rapporto di fiducia.

Che le cosiddette ecoballe - sono molto balle e poco eco - vengano trasferite da Giugliano ad Acerra e che Acerra diventi il ricettacolo di tutto è un fatto che non può stare né in cielo né in terra. terra. Acerra si è fatta carico e deve farsi carico - lo dico chiaramente - del termovalorizzatore, il quale deve partire. Ma Acerra ha anche bisogno da oggi, e non da domani, di una di una operazione di bonifica seria, vera. I filmati che abbiamo visto, che sono reali, oltre a danneggiare l'economia della Campania e dell'intero hanno danneggiato la salute dei cittadini, e non è colpa del termovalorizzatore. È colpa di tutta quella operazione nefanda, gestita in buona parte dalla malavita, che avviene in quei terreni a confine. le dichiarazioni del sindaco di Acerra con le quali dà la colpa ai pastori che sbagliano nel portare a pascolare le pecore, perché un cippo in mezzo a un campo divide l'area buona da quella cattiva. Delle discariche già previste ho parlato. Bisogna che lavoriamo e che diamo i poteri veri al commissario per individuare nuovi siti. Non possono essere - l'ho già detto - sempre le solite aree ad essere sacramentate. Bisogna avviare una operazione di sanificazione del territorio campano, dove si trovano tra i 1.400 e i 1.500 siti abusivi censiti, e non so quanti siano quelli non censiti.

determinante di un ciclo completo e moderno per il trattamento dei rifiuti. Ma, se la raccolta differenziata è rimasta al palo fino ad oggi, non può nemmeno essere questa la soluzione dell'emergenza.

avvenuto in tante città in anni passati, un processo che deve passare anche attraverso le amministrazioni e la classe politica campana, la quale deve avere il coraggio di guidare il cambiamento nella propria Regione.

illecita? Utilizziamo seriamente i militari.

analoghi a quelli della magistratura. Credo che la suddetta Commissione debba intervenire ancora di più sul territorio presidiando e costringendo magistratura e amministrazioni locali

Presidente, prima di iniziare il mio intervento devo fare una confessione. Come uomo del Nord e socio fondatore della Lega,

che Napoli mi sia rimasta nel cuore come città e le immagini che la televisione trasmette tutti i giorni mi hanno fortemente turbato. Volendo dare un titolo politico alla crisi del problema immondizia della Campania si potrebbe parlare del grande fallimento dello Stato centralista che di tutto si vuole interessare e nulla riesce a combinare. Anzi, dopo aver ascoltato il ministro Bonino ieri in Commissione ho capito che oltre alla beffa ora arriverà il danno che culminerà in una gravosa sanzione economica da parte dell'Europa nei confronti dell'Italia. Spontaneamente viene da dire "bravi, 7 più" a quelli che irresponsabilmente si sono adoperati per arrivare a tali risultati. mi sono chiesto come mai gli istituti preposti al controllo della cosa pubblica non hanno fatto sentire a tempo la propria voce. Così ho fatto un po' come San Tommaso. Un mese fa sono andato a Napoli per rendermi conto personalmente di come la città vivequesto dramma.

Il mio sconforto, dopo questo viaggio, è ancora maggiore. Da sempre sono animato da quel fuoco federalista che vive in me e che lavora in un modo che la politica, in particolar modo amministrativa, non sia né di destra né di sinistra ma al servizio completo della società per il miglioramento della qualità della vita di tutti. Il vero federalista vive il suo fare politica come la massima espressione della carità. Le cose, invece, sono andate e continueranno ad andare esattamente al contrario proprio perché il modello ed il pensiero federalista è così lontano e l'informazione di Stato non ha fatto nulla per diffonderlo. Anche quella del nostro Paese è una informazione-spazzatura. Non mi è mai capitato di vedere in televisione il pensiero di padri del federalismo come Cattaneo, Rosmini o Gioberti, un confronto di come si svolge la vita amministrativa, ad esempio, presso la Confederazione svizzera o la Repubblica federale tedesca: da sempre si dipinge il mio movimento - ed è quello che fortemente mi preoccupa - come razzista, egoista, xenofobo mentre siamo esattamente all'opposto, e ve lo dice uno che la Lega l'ha fondata. È chiaro che chi semina vento non può che raccogliere tempesta. Non dimentichiamo che uno dei princìpi fondamentali del federalismo è di ragionare uno per tutti e tutto per uno. In una logica federalista la Regione Campania avrebbe dovuto affrontare il problema immondizia il giorno dopo che la sua cittadinanza ne avesse avuto bisogno. Se il suo territorio non è adeguato doveva scattare da subito un progetto di sussidiarietà con le Regioni limitrofe, con un piano di lavoro, di interscambio sussidiario per cui io ti do e tu mi dai, per ovviare a tale necessità. Sono pensieri e progetti così nobili che l'oscurantismo centralista farà di tutto per non far riconoscere,

Molte di loro sono poste in uno Stato centralista; sono dei carrozzoni costosi che producono inefficienze paurose. Ecco perché i conti del Paese Italia non tornano e non torneranno mai.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, l'emergenza rifiuti in Campania è un disastro ambientale, economico e di immagine senza precedenti. È la diretta conseguenza di anni di errori, omissioni e malgoverno. Una montagna di "monnezza" che non solo ha ricoperto le strade della città campana, ma ha già sommerso cinque commissari straordinari e bruciato miliardi di euro. È vero, colleghi: la criminalità organizzata ha sempre fatto la parte del leone in quell'area del Paese, infiltrandosi nel settore dei rifiuti con lo smaltimento illegale e, comunque, in tutti i sistemi economici. Ma quello che salta subito agli occhi sono le responsabilità di chi governa ed ha governato in questi anni; l'intreccio di interessi politico-affaristici, gli sprechi di denaro, le assunzioni clientelari di massa; responsabilità che hanno nomi e cognomi, a cominciare dal sindaco Iervolino fino al presidente Bassolino che da 15 anni è sovrano incontrastato prima di Napoli e poi dell'intera Campania, senza trascurare il fatto che fino a poco tempo fa era persino commissario straordinario per l'emergenza rifiuti. E come non citare in questa partita il ministro dell'ambiente Pecoraro Scanio, incapace di gestire in questi anni l'emergenza rifiuti che era pronta a scoppiare, ma nel contempo deciso, in nome di una paventata salvaguardia ambientale, ad osteggiare qualsiasi soluzione al problema, dalla individuazione di nuovi siti per lo stoccaggio sino alla realizzazione dei termovalorizzatori. E che dire del presidente Prodi, che non è stato in grado di gestire prontamente l'emergenza campana, di prendere decisioni concrete ed efficaci salvo poi "sbottare" per la mancanza di solidarietà dalle altre Regioni. È davvero disarmante la calma e la tranquillità che accompagnano il presidente Prodi di fronte alle gravi responsabilità delle amministrazioni campane; di fronte al disastro di questi 15 anni di amministrazione di sinistra; d'altronde, si sa che qualcuno «tiene famiglia» (qui a Roma e, in modo particolare, qui al Senato) e di questi tempi è meglio forse non tirare troppo la corda. corda. È altrettanto sorprendente il fatto che, tra i colleghi del centro-sinistra, nessuno abbia avuto la fermezza ed il coraggio di chiedere ed ottenere le dimissioni degli artefici compiacenti dello scempio attuale e di quelli passati: tutti ben saldi ed incollati al proprio centro di potere. Tutti stanno zitti, anche quando a livello internazionale andava in onda lo spettacolo di una città sommersa di cumuli di rifiuti; anche quando in gioco non c'è soltanto l'immagine di Napoli e della Campania, ma dell'Italia intera. Presidente Prodi, lei chiede solidarietà e definisce una vergogna nazionale il rifiuto di alcune Regioni di accettare parte dei rifiuti campani. Vede, di fronte all'immobilismo del Governo e alla faccia tosta con cui si sta affrontando questa emergenza, i Governatori delle Regioni dovrebbero ben riflettere prima di accettare tacitamente tonnellate di rifiuti senza nessun controllo. Colleghi, come ben sapete io sono sardo e la Sardegna, per esclusiva volontà del presidente Soru, è stata la prima Regione a ricevere parte dei rifiuti campani con una azione politica e mediatica condotta in solitaria e - soprattutto - senza alcuna concertazione, che ha suscitato le ire e le proteste di coloro che si sono visti recapitare a domicilio, a due passi da casa, una nave carica di rifiuti senza neanche poter dire una parola. Presidente,colleghi, e concludo, è incredibile che davanti ad una situazione come quella campana, vergogna nazionale ed internazionale, sia consentito ai responsabili di questo disastro di restare al loro posto, ostinatamente e sfacciatamente, e ancor più con il *placet* di questo Governo. Signor Presidente,colleghi, e concludo davvero, le immagini di una parte del Paese sommersa dai rifiuti, le immagini dei ragazzi impossibilitati ad entrare a scuola l'esasperazione della gente dovrebbero portare tutti, unitariamente, a chiedere le dimissioni di chi ha delle responsabilità, cioè le dimissioni del presidente Bassolino. PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liotta. Ne ha facoltà. signor Ministro, onorevoli senatori, la vicenda campana evidenzia responsabilità molto gravi delle amministrazioni locali e il sostanziale fallimento dei pur necessari strumenti straordinari adottati. Oggi, davanti al disastro sociale e ambientale sotto gli occhi di tutti, non vorremmo che sull'altare dell'emergenza venissero sacrificati princìpi sacrosanti di salvaguardia ambientale e di salute dei cittadini. Le Regioni sono chiamate alla solidarietà nazionale, ma già vi è chi interpreta in senso strumentale il concetto di solidarietà. non è stata la prima e unica Regione ad aver aperto le braccia alla spazzatura campana in segno di solidarietà. Non per la prima volta la Sicilia è una delle prime Regioni che ha aperto le braccia alla spazzatura campana: già l'anno scorso ricorderete che, nell'acutizzarsi della crisi e dell'emergenza campana, la Sicilia accolse navi di rifiuti provenienti dalla Campania e poi lo stesso ambiente di centro-destra si accoglieva la spazzatura e chi, invece, ostacolava l'ingresso delle navi nel porto di Catania. In Sicilia oggi si sta verificando uno sporco baratto tra l'accoglimento della spazzatura campana e la realizzazione dei quattro termovalorizzatori previsti dal piano regionale dei rifiuti. La Sicilia è stata commissariata per l'emergenza rifiuti per circa cinque anni e il prodotto di tale commissariamento, oltre alla dissipazione di ingenti risorse finanziarie da parte della struttura commissariale, è stato un piano regionale dei rifiuti centrato essenzialmente sugli inceneritori, quindi sulla scorciatoia che, saltando tutti i passaggi previsti dalla legislazione nazionale ed europea (la riduzione, il riuso, la raccolta differenziata),

A quegli imbonitori dei termovalorizzatori che volessero contrabbandarci questa idea negatrice del principio di conservazione della massa, ricorderemo che essi non non distruggono massa, ma semplicemente la trasformano e la redistribuiscono: 100 chili di spazzatura entrano dentro gli inceneritori e 100 chili di spazzatura escono da ogni termovalorizzatore, da ogni inceneritore. Semplicemente, prima erano tutti allo stato solido e, dopo, 70 chili sono allo stato aeriforme e 30 in forma di polveri ancora allo stato solido, quindi necessitano di essere stoccati in discariche speciali, perché sono classificati come rifiuti

Noi siamo abituati a parlare di ecomafie riferendoci essenzialmente alla criminalità delle discariche e diciamo: facciamo i termovalorizzatori, perché se saltiamo tutti i passaggi del ciclo integrato dei rifiuti (se saltiamo la riduzione, il riuso il riuso e la raccolta differenziata, perché i cittadini non la vogliono fare), non rimane altro che la termovalorizzazione, così non avremo la difficoltà di contrastare l'inquinamento mafioso all'interno della realizzazione delle discariche. Ebbene, in Sicilia su quattro termovalorizzatori, la presenza la presenza delle infiltrazioni mafiose è già stata segnalata dalla magistratura almeno in uno dei quattro raggruppamenti temporanei di imprese che si sono messe insieme per costruire i quattro impianti.

quattro termovalorizzatori in quattro territori non scelti dalla Regione siciliana. Mi chiedo cosa dovrebbe fare un'amministrazione che, pur volendo procedere fino al passaggio finale del ciclo integrato dei rifiuti, si atteggiasse a una programmazione sul proprio territorio. Verificherebbe gli ambienti anche sotto il profilo urbanistico e della vocazione industriale in cui possono essere inseriti impianti che possono includersi a valle del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti. Ebbene, sapete come sono stati scelti i quattro siti dei quattro impianti siciliani? Sono stati scelti dai quattro raggruppamenti dai quattro raggruppamenti temporanei di impresa che hanno avuto affidata la concessione della Regione siciliana. Non è la Regione che ha programmato sul proprio territorio la distribuzione degli impianti: le ditte che hanno avuto l'affidamento hanno scelto dove costruire gli impianti. Uno di questi casi lo il presidente Matteoli, perché ha avuto occasione di partecipare in quel territorio a un'affollatissima assemblea qualche anno fa, quando si è cercato di calare questo impianto di termovalorizzazione in quel territorio. In uno di questi territori l'impianto di termovalorizzazione è previsto all'interno di un sito di interesse comunitario, a 200 metri dall'asta fluviale più importante della Sicilia. La Sicilia non ha molti fiumi; la Sicilia è presidio è presidio ambientale contro la desertificazione e possiede pochissime aste fluviali. Nel territorio di quell'unica grande asta fluviale, che alimenta l'elemento ambientale di maggiore ricchezza economica di quella Regione (ossia la piana di Catania, dove si produce il 60 per cento delle arance che si mangiano in Italia), dentro un sito

europee per l'affidamento delle concessioni. Oggi, sull'onda dell'emergenza, il Governo dichiara che i quattro termovalorizzatori in Sicilia verranno realizzati. Il quadro normativo attuale che abbiamo scritto sulla finanziaria non consente la concessione dei contributi CIP6 ai quattro termovalorizzatori siciliani. Il Governo sappia che non consentiremo aggiramenti di quella normativa e che su di essa bisogna attestarsi. I quattro termovalorizzatori siciliani sono un insulto all'ambiente e all'economia della Sicilia. Noi non vorremmo che l'emergenza pagasse Cuffaro e che il prezzo debba essere pagato dai cittadini. Se Cuffaro accoglie poche migliaia di tonnellate di rifiuti e lo scambio iniquo che intende fare questo Governo è quello di poche migliaia di tonnellate di rifiuti in cambio della costruzione dei quattro termovalorizzatori, il Governo sappia che ci troverà come ostacolo su questo percorso.

la vicenda dell'emergenza rifiuti in Campania, i cui effetti sono ormai sotto gli occhi di tutto il mondo, tra i tanti guasti che ha provocato certamente potrà annoverare anche le profonde modifiche che ha comportato nel lessico, nel significato delle parole. Continuiamo a definire emergenza una vicenda che l'11 febbraio prossimo compirà il suo quattordicesimo anno. In quale campo delle attività umane non si sarebbe trasformato almeno il vocabolo? In medicina, alla parola "crisi" si fa subentrare la definizione di "stato di male" quando una condizione si protrae per alcune ore; anni avrebbero dovuto consigliare almeno questo. Pensiamo anche che ad un certo punto si è utilizzata una serie di sistemi che servono per affrontare le catastrofi naturali. Si è utilizzato il sistema della protezione civile, si è invocata la solidarietà nazionale e negli ultimi giorni si è evocata l'immagine di Firenze e degli angeli che accorrevano da tutto il mondo ad aiutare la città inondata dall'esondazione dell'Arno. Vi chiedo se è possibile utilizzare questo tipo di categorie per una situazione come quella della Campania. Si può definire imprevista la produzione dei rifiuti e la conseguente necessità di provvedere al loro smaltimento, quando si è in grado di prevedere la quantità dei rifiuti che saranno prodotti e addirittura la loro composizione percentuale

deve guardare alla propria storia - si sono nel tempo verificate emergenze rifiuti: nei primi anni Novanta in Toscana e verso la metà degli anni Novanta in Lombardia.

lì è stata colta l'occasione per incrementare la raccolta differenziata, realizzare impianti e predisporre la chiusura del ciclo. Oggi quelle Regioni non avvertono più la condizione emergenziale. In Campania tutto questo non è avvenuto e paradossalmente l'emergenza ha provocato una grave deresponsabilizzazione delle istituzioni e delle amministrazioni locali, spesso tentate esse stesse di farsi capofila delle proteste contro qualsivoglia impianto si intendesse realizzare, fosse esso discarica, impianto di compostaggio o addirittura stazione di trasferenza. Ci si è opposti praticamente a tutto e spesso in prima fila, a fianco a politici - ricordo Sottosegretari in carica e segretari nazionali di partito

Questa è la testimonianza che lì qualcosa si è rotto e che non debba sfuggire la gravità della situazione lo dimostra anche il fatto che, diversamente dalle ultime volte,

parte vi è lo smaltimento illecito dei rifiuti industriali - spesso tossici - in ampie aree del territorio campano, soprattutto casertano e napoletano, che costituisce un drammatico fenomeno che ha visto l'intrecciarsi di interessi illeciti tra le imprese ed una camorra che ha offerto sistemi economici di smaltimento. Questo chiama anche il Parlamento alla sua responsabilità,

un'attività di indagine penetrante e capace, oggi non avremmo nei fatti armi, perché i reati contro l'ambiente sono, per la stragrande maggioranza, contravvenzionali, per cui spesso vengono puniti con un'ammenda e hanno tempi di prescrizione talmente irrisori che chiunque sa di poter commettere un reato senza correre il rischio di scontare alcuna pena.

Perché questo è il motivo per cui si utilizza l'Esercito: togliere una delle principali fonti di finanziamento ai sistemi illeciti che sono dedicati al trasporto dei rifiuti. Si utilizzano il Genio e l'Esercito per rompere il circuito che porta grandi risorse nelle casse di ecocriminali non sempre camorristi, qualche volta anche con il colletto bianco. La Commissione bicamerale ha messo per iscritto (e noi siamo d'accordo con quella impostazione) una via di uscita, che prevede: un accordo istituzionale di programma tra Governo e istituzioni locali che le accompagni all'uscita dall'emergenza; lo scioglimento della struttura commissariale, spesso infiltrata anch'essa dalla malavita; l'individuazione, da subito, di un numero congruo di siti da adibire a discariche di soccorso o a piazzole di stoccaggio; della solidarietà nazionale che sarà più facile conseguire quando la Campania avrà dimostrato di avere un progetto chiaro per uscire da quella emergenza; l'accelerazione, da subito, del completamento di Acerra e degli altri impianti che possono consentire un ciclo integrato dei rifiuti. La Campania non è terra persa, perché se a Salerno e nella sua provincia molte comunità sono in grado di raggiungere risultati brillanti vuol dire che ci vuole solo l'azione della politica, della buona politica, perché i cittadini, quando sollecitati, sono in grado di offrire la collaborazione necessaria. C'è bisogno di uno sforzo della Nazione, ma il primo pezzo di Paese che si deve muovere è certamente la Campania. nuova finestra"). Ho il piacere di salutare tra il pubblico che sta assistendo a questa seduta le allieve e gli allievi della scuola media «G. Pascoli» di Benevento.

Signor Presidente, al termine di un dibattito così ampio, mi limito a sottolineare alcune questioni di carattere generale. La prima credo riguardi questo ciclo negativo, che ormai si avvita da oltre quattordici anni, nella situazione della gestione dei rifiuti della Campania, tra straordinarietà della gestione ed emergenza, e fra emergenza e straordinarietà. Siamo partiti da situazioni emergenziali che hanno richiesto interventi straordinari. Il continuare, il perpetuarsi di interventi straordinari negli anni ha, a mio avviso, mantenuto e rigenerato emergenza. Questo circuito negativo noi lo vogliamo interrompere e ribadisco che è intenzione del Governo ritornare al più presto ad una gestione ordinaria della questione dei rifiuti nella regione Campania, ribadendo quindi che al commissario De Gennaro il Governo ha dato un incarico che si esaurisse nei centoventi giorni, che riteniamo indispensabili per uscire dalla fase più acuta dell'emergenza. Ritornare all'ordinarietà vuol dire ricominciare in maniera visibile ad avere un'assunzione di responsabilità forte delle istituzioni locali campane, una assunzione che deve avvenire a partire anche dalle scelte che riguarderanno la fase più acuta dei prossimi giorni. A questa assunzione di responsabilità delle istituzioni non deve mancare un impegno civico dei cittadini campani. Ho accennato, nella mia relazione, all'idea del commissario di avviare una forma straordinaria di alleggerimento della produzione di rifiuti o, per meglio dire, della messa in strada dei rifiuti, in particolare di rifiuti che possono avere una destinazione di riciclo (penso alla carta e al vetro) per alleggerire anche le dimensioni del problema. Alla fine di un percorso di questo tipo credo potremo più utilmente fare riferimento all'impegno ed alla solidarietà delle altre Regioni.

questa occasione per demonizzare il rifiuto ed il ciclo di smaltimento perché, come veniva ricordato prima, anche altre realtà hanno vissuto momenti di emergenza e non è che l'intero sistema nazionale sia privo di punti di criticità. rifiuti, evidentemente, va fatta un'azione preventiva; produrne meno è l'elemento di lungo periodo che tutti dobbiamo privilegiare, ma sappiamo anche che i rifiuti vanno smaltiti e che è possibile farlo in sicurezza, con tecnologie e sistemi adeguati. La solidarietà sarà importante ma è del tutto evidente che il grosso del problema dovrà essere risolto in Campania. Ribadisco che

Da più di due mesi i ministri Bersani e Pecoraro Scanio hanno in mano il piano del professor Contò che sviluppa l'esperienza fatta a Treviso con una raccolta differenziata spinta ed il relativo recupero e riciclaggio di rifiuti urbani. Potrà non piacere che a Treviso ci sia una certa colorazione politica ma non mi pare il caso di fermarci a questi distinguo. Vorrei sapere perché di questo non si parla. Qui il ministro Santagata, lasciato solo stamattina dal Governo - ma non è che l'Aula brilli per un maggiore interesse - ci propone di avviare in tempi medi un piano per la raccolta differenziata. Dal febbraio 2007 è a disposizione la relazione del professor Giovan Battista de' Medici che individua le aree vocate alla realizzazione delle discariche. Il Governo, invece, stamattina dichiara che è ancora prevista la soluzione Pianura, che è criminale.

Già è stato spiegato in altri interventi che non inceneriscono un bel niente e tanto meno termovalorizzano, visto che esce il 10 per cento dell'energia introdotta. Ma è dal IV secolo a.C. che e nulla si distrugge. Finisce che poi ce lo respiriamo o ce lo mangiamo, tant'è che non è più possibile in Campania, nelle province di Napoli, Salerno e Caserta, tenere le pecore al pascolo perché immetterebbero nel ciclo animale e alimentare sostanze tossiche dannose per l'organismo. Vi sono alcune tabelle europee che stabiliscono quanto costa al sistema sanitario nazionale la realizzazione dei cosiddetti termovalorizzatori. Invito, quindi, il nuovo partito americano

lodo la sua licenza di concedere più tempo e quindi ne approfitterò, pur tentando di restare nei tre minuti Ho sufficiente conoscenza della Costituzione per sapere che il Governo in Aula si fa rappresentare da chi decide, però mi consenta una valutazione di carattere politico. La vergogna dei rifiuti che seppellisce la Campania non credo c'entri molto con l'attuazione del programma di Governo, per cui ci saremmo aspettati, in questa sede, la presenza del Ministro dell'ambiente o

una città che pare rassegnata e messa in ginocchio al punto che i cittadini di quella terra devono pagare ancora la tassa sui rifiuti, nonostante questo servizio non sia garantito. Signor Presidente, avrei voluto la presenza di un Ministro competente sul tema anche per chiedere conto di una preoccupazione che abbiamo espresso anche a nome del movimento politico La Destra. Ma davvero il problema dei rifiuti, come ha detto il Presidente del Consiglio, è una questione di immagine dell'Italia nel mondo? Non è più importante forse la salute da garantire ai cittadini di Pianura? Credo che su queste questioni avremmo dovuto confrontarci in maniera seria e certo non mancherà l'occasione della discussione quando si parlerà

Quando sono stato a Napoli qualcuno ha tentato di fare lo spiritoso, risalendo alle responsabilità che si perdono nel tempo, risalenti a tredici anni fa. Antonio Rastrelli, un galantuomo di antico stampo, varò un piano di rifiuti e poi fu cacciato da quella mala politica che, guarda caso, in queste ore è messa sotto inchiesta dalla magistratura campana. Oggi si torna ad un piano rifiuti che prevede gli stessi impianti indicati nel piano Rastrelli, mai attuato dalle maggioranze che si sono alternate. Credo che il Parlamento - e mi avvio a concludere, signor Presidente, rinunciando alla licenza che volevo prendermi

per dare attuazione, per la prima volta nella storia della Repubblica, all'articolo 126 della Costituzione. È una grande questione legata anche la sicurezza nazionale. Il Parlamento ha il dovere di rappresentare le istanze dei cittadini campani. Voteremo i documenti che vanno nella direzione di conferire un segnale chiaro e di una politica che finalmente decide. Signor Presidente, le tragiche immagini, che vediamo in questi giorni, stanno creando un vero e proprio danno strutturale e - direi - antropologico alla Regione Campania. Il danno non solo di immagine, ma anche alla capacità di attrarre turismo ed investimenti non l'ha mandato Dio. Dio manda gli uragani e i terremoti; l'immondizia che si accumula per quattordici anni, creando quello che efficacemente è stato definito l'ossimoro emergenza, la mandano gli uomini, le scelte sbagliate o le non scelte degli uomini. In questo caso le responsabilità risalgono all'intera filiera istituzionale campana

per la tutela della pubblica amministrazione. Veniva citato il livello delle tecnologie scelte. Il secondo errore è stato quello di non decidere in maniera risoluta di dotare la Campania di un ciclo industriale di rifiuti che, partendo da alti livelli di raccolta differenziata, arrivasse attraverso impianti intermedi ad avere gli impianti di smaltimento finale. Sottolineo il combinato disposto tra alti livelli di differenziata ed impianti di smaltimento finale che, dovunque, nelle aree più avanzate vanno insieme.

è verificata la crescita di un sistema di intermediazione, di un vero e proprio reticolo clientelare, di consorzi e di un commissariato che aumenta a dismisura. un vero e proprio sistema di potere che, ogni volta che si profilava la possibilità di uscire dall'emergenza, si è opposto con ostruzionismo e anche peggio all'uscita dall'emergenza stessa. Di straordinario, dunque, abbiamo avuto solamente la burocrazia, l'intermediazione e la clientela, non i poteri di decidere. Anche il Governo ha le sue responsabilità, ministro Santagata. Già da giugno, infatti, la Commissione d'inchiesta sui rifiuti aveva indicato la soluzione: quando gli enti locali non sono in grado di decidere, nei Paesi civili ci sono i poteri sostitutivi del Governo, anche immediati. Anche nell'America federale, lì dove nella Louisiana dopo l'uragano Katrina il governatore locale non fu capace di risolvere i problemi, fu sostituito dallo Stato centrale. Ora, con l'ultima ordinanza del Governo, abbiamo delle interessanti novità. Sottolineo, però, ministro Santagata, quelle che ritengo siano - e qui rappresento tutta la Commissione rifiuti -- le azioni da fare e le modalità da seguire. smantellare immediatamente i consorzi. Nell'ordinanza è scritto semplicemente che con successivo provvedimento sarà fatto; va fatto immediatamente. smantellare immediatamente l'intera struttura commissariale, facendo rientrare alle amministrazioni di appartenenza tutta la burocrazia distaccata con indennità, chiudendo le consulenze e azzerando tutti i costi per la pubblica amministrazione. necessario far sì, ministro Santagata, che per i centoventi giorni restanti, prima di tornare ai poteri ordinari, il prefetto De Gennaro più che un commissario sia un vero e proprio soggetto attuatore di decisioni prese da un accordo istituzionale.

fino allo scioglimento degli enti locali inadempienti, temo che il prefetto De Gennaro non sia in grado di fare meglio di quanto fatto da suoi autorevoli predecessori. Quindi, per cortesia, è sufficiente elaborare

quindi la fine del commissariato, un accordo istituzionale di accompagnamento e finalmente, nelle giuste sedi, un ciclo industriale dei rifiuti, con una raccolta differenziata adeguata, effettuata da chi ordinariamente deve occuparsene, e impianti di smaltimento finale, che sono i termovalorizzatori o le migliori tecnologie disponibili per l'obiettivo dello smaltimento finale. Signor Presidente, signor Ministro, siamo di fronte non ad un'emergenza, ma ad una tragedia. Il nostro Paese civile e democratico sta per perdere un'area culturalmente, sta per perdere un'area culturalmente, geograficamente e storicamente importante. Quando il 90 per cento dei ragazzi non può andare a scuola, è una situazione di tragedia. Chiedo per cortesia al Governo di andare oltre l'ordinanza e di convocare immediatamente il tavolo istituzionale per le decisioni necessarie. Passata questa fase di emergenza, poi si parlerà anche della responsabilità degli enti locali. Chi ha sbagliato pagherà fino in fondo e i cittadini giudicheranno con le elezioni, anche anticipate, se è il caso.

decine di quintali di rifiuti solidi urbani stazionano ormai da settimane nelle strade della Campania ed oltre 100.000 studenti continuano a non andare a scuola. Possiamo far finta di niente, rispetto ad un serio rischio di patologie infettive, trasformatosi ormai, giorno dopo giorno, in una triste certezza? Possiamo far finta di niente rispetto ad una emergenza che, attraverso forme diverse, si prolunga ormai da anni, deteriorando ed inquinando la stessa immagine del nostro Paese all'estero? Possiamo far finta di niente di fronte ai picchetti, alle polemiche spontanee e non strumentali di tanta gente di Pianura, che dopo quarantuno chiede giustamente che i rifiuti vengano portati altrove, che si sviluppi finalmente un serio biomonitoraggio, in grado di far comprendere i danni reali, effettivi realizzatisi sulla popolazione residente? Possiamo infine far finta di niente rispetto ad una emergenza che si intreccia ormai da anni con la criminalità organizzata e che ha fatto muovere inutilmente cifre di milioni e milioni di euro? Mentre spuntano questi interrogativi, cari colleghi, emerge il problema più drammatico e vero. Appare ormai certo, come è stato testimoniato anche ieri da «Il Sole 24 ORE», che in Campania sono stati sepolti illegalmente quintali di rifiuti tossici e nocivi, oltre il 35 per cento dei rifiuti tossici e nocivi che sono stati prodotti nel nostro Paese. È questo, Presidente, il vero, grande disastro ambientale della Campania. È questa, al di là dei rifiuti solidi urbani, la spia più inquietante che produce ormai gravissimi danni ambientali, ma anche terribili danni sull'intero territorio.

Se il «Lancet oncology», una delle più prestigiose riviste scientifiche internazionali, lancia segnali inquietanti sul triangolo Nola, Acerra e Marigliano, se l'Organizzazione mondiale della sanità conferma la gravità della situazione sanitaria in Campania, se il problema riguarda la contaminazione di alimenti, di animali e quindi di persone, dobbiamo necessariamente prepararci ad anni difficili e complessi.

e ci meraviglia la posizione di alcune forze politiche, come quelle legate al ministro Di Pietro, che in Campania chiedono lo scioglimento del Consiglio e altrove si pronunciano per la sua permanenza. Non c'è stato in tal senso tal senso il soprassalto di orgoglio che avevamo auspicato e questo ci costringe a non poter firmare la risoluzione della maggioranza e a richiedere a quest'Assemblea l'assunzione di un forte atto di responsabilità nei confronti della Regione Campania.

Signor Presidente, l'Unione Democratica per i Consumatori ritiene che anche in quest'Aula del Senato sia giunto il momento di fare chiarezza su una vicenda torbida ed inquietante contrassegnata fin qui da una sola consegna per tutti: l'obbligo di un silenzio che, mai come in questo caso, diventa insopportabilmente colpevole perché evita di ricostruire e di attribuire le responsabilità. anni abbiamo dovuto registrare un fallimento che appare inequivocabilmente riconducibile sia ai livelli regionali - irresponsabili ed incapaci quando non collusi ed interessati, giunti fino al punto di fare dell'emergenza rifiuti uno strumento originale di intermediazione clientelare, rimodulando uno schema già utilizzato negativamente nel *post*-terremoto sia ai livelli politici nazionali, più interessati a coprire le inettitudini ed i disastri locali, fino al punto di non affrontare la questione dell'assenza di un ciclo integrato dei rifiuti in Campania e dei relativi impianti industriali, lasciandola così incancrenire tanto che oggi, dopo i disordini di Napoli, dopo i roghi, le occupazioni e le violenze, è diventata un problema sociale, gestionale ed igienico-sanitario difficilmente risolvibile. La gestione dei rifiuti in Campania è diventata l'emblema di un fallimento campano e nazionale che anche l'Europa ci contesta. Il ministro Emma Bonino, ascoltata ieri in Commissione 14a al Senato, ha confermato che la Commissione europea deciderà il prossimo 30 gennaio

Il fallimento che abbiamo di fronte ci obbliga moralmente e politicamente a scelte chiare e decise, senza voler assolutamente ricercare unanimismi di facciata che, nel tentativo di accontentare tutti, finiscono con il perdere di vista il reale obiettivo. Occorre innanzitutto tradurre in realtà le promesse, cominciando dall'immediato scioglimento di strutture clientelari inutili e dannose quali i consorzi. È necessario poi recuperare l'importante contributo offerto dalla Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, che ha più volte suggerito la strada dell'accordo di programma, ritenendo decisivo che non si creino ulteriori sovrastrutture e che Governo, Regione, Province e Comuni capoluogo vengano chiamati ad individuare la strategia necessaria per assicurare alla Campania una gestione dei rifiuti finalmente efficiente, prevedendo immediatamente incisivi poteri sostitutivi nei confronti di quegli enti locali che non avranno saputo far fronte alle loro responsabilità. Se la malattia è grave, la cura dev'essere necessariamente energica. Ho l'impressione che la terapia proposta sia ancora troppo debole ed inefficace. Occorre fare di più. Siamo pronti ad assumerci la nostra parte di responsabilità. Ecco perché non abbiamo sottoscritto la risoluzione della maggioranza, preferendo invece condividere la proposta Barbieri, anche se leggermente modificata. *(Applausi

verso l'attuale governo regionale e i governi a guida Unione o a guida centro-sinistra. Facciamo, infatti, una valutazione che scaturisce dagli anni trascorsi da quando la nostra coalizione ha assunto il governo in Regione e in tanti enti locali. Noi pensiamo chenon si possa più restare in questa fase in cui si critica ciò che è stato fatto o non è stato fatto da chi ha preceduto la nostra coalizione.

I nostri consiglieri regionali hanno anche sottoscritto, per primi, una mozione di sfiducia che non ha trovato il numero di firme sufficiente per essere discussa. La nostra posizione, così netta, non ci porterà mai comunque ad essere strumento nelle mani dell'altra coalizione, che in quanto a responsabilità ha anch'essa da farsi perdonare diverse cose.

auspichi una svolta politica e gestionale delle istituzioni locali attraverso un profondo rinnovamento delle amministrazioni. La chiave di volta è ricostruire un rapporto di fiducia con gli elettori, che presuppone anche un cambio di persone alla guida dei nostri enti locali. Credo che la nostra maggioranza si stia seriamente avviando a prendere in considerazione questa ipotesi.

In sostanza, ha inteso dire: non occupiamoci del passato, ma guardiamo al presente e rimbocchiamoci le maniche. Ha poi concluso ricordando che senza l'adesione e l'impegno delle popolazioni locali non si va da nessuna parte. Certamente, è così. Ebbene, signor Ministro, noi cogliamo una contraddizione e un punto di debolezza. La crisi odierna a Napoli e in Campania non è soltanto un drammatico danno di immagine a livello mondiale, è soprattutto una devastante crisi di credibilità della politica e delle istituzioni, che rischia addirittura di non potersi limitare al livello locale. I tumulti, le proteste e i blocchi stradali non sono soltanto il frutto di pochi facinorosi, magari sobillati dalla camorra. Se così fosse, basterebbero gli interventi in chiave di tutela dell'ordine pubblico a risolvere il tutto. Invece, abbiamo il rifiuto delle popolazioni locali di affidarsi alle istituzioni. Prevale la sfiducia, il rigetto. Se non si supera questo stato di cose non si può vedere la fine del tunnel. Le istituzioni in Campania hanno l'autorità formale, i poteri, ma hanno perso qualsiasi autorevolezza. E nello spazio che divide appunto la forma, cioè l'autorità, dalla sostanza, che è l'autorevolezza, si colloca la crisi. Questa distanza viene appunto dalla storia pregressa, dal lungo susseguirsi di errori, di scelte clientelari, di malapolitica e malamministrazione. Da anni vediamo sui mezzi di comunicazione di massa inchieste devastanti. Spesso ci siamo chiesti come mai la magistratura non prendesse o non portasse avanti con la decisione necessaria le opportune iniziative. Poche, pochissime le voci nella politica regionale e locale - tra queste la mia e quella del senatore Sodano - che da tempo hanno chiesto un cambiamento radicale. Abbiamo assistito per anni ad una politica sorda; ad un drammatico fallimento del ceto politico e di governo, di una intera classe dirigente che ha accomunato tutte le forze politiche, non certo solo questa o quella; a una società civile torpida; ad istituzioni lente, distratte, disattente. Non si capisce e non si affronta la crisi di oggi senza tener conto di questo passato. Non si recupera credibilità se non ci si pone la domanda su chi risponde di cosa. È stupefacente che tutto accada senza che nessuno se ne assuma con chiarezza la responsabilità. È stupefacente che i cittadini napoletani e campani paghino - oltre che una tassa sui rifiuti, che nella situazione data è una sorta di estorsione legale, una gabella medievale - un prezzo altissimo in termini di salute, e che tutti facciano finta di niente. Io stesso ho ricordato anche in questa Aula come addirittura l'aspettativa di vita dei cittadini napoletani e campani sia più breve di quella dei cittadini di altre Regioni. E cosa è accaduto? Esattamente nulla. Non si recupera credibilità senza una rottura con il passato, senza una evidente ed indiscutibile discontinuità. Non possono rimanere in piedi le strutture come i consorzi e non solo, nelle quali malapolitica e malagestione hanno trovato un favorevole terreno di cultura. Non può la gestione del problema rifiuti rimanere nelle mani delle stesse persone che hanno concorso a determinare il disastro di oggi. Quelle persone possono mantenere l'autorità formale, ma di certo non potranno riguadagnare autorevolezza. Discontinuità dunque, rottura, facce nuove di persone che non siano gravate dal peso di compromessi e collusioni. Andare avanti su questa strada con coraggio, senza calcoli politicisti; tagliare corto con clientele, superfetazioni burocratiche, interessi inconfessabili e collusioni piccole e grandi. Questo non è un furore giustizialista, ma la convinzione che solo così si avvia la soluzione della crisi, solo così si riguadagna quella credibilità che è il passo necessario

Abbiamo di fronte un tempo non breve, che sarà comunque di crisi. È bene che ci rendiamo conto di questo. Le soluzioni strutturali non potranno essere adottate, perfezionate, completate e messe in opera nell'arco di qualche settimana o persino di qualche mese. Quindi, se è così, se il tempo che abbiamo comunque davanti sarà di emergenza perdurante, di durata non breve, dobbiamo capire che non è possibile affrontarlo solo con le scarpe chiodate di poteri speciali.

anche in Aula, anche nelle comunicazioni del Governo, è stata definita come indispensabile. Con queste motivazioni, signor Presidente, noi voteremo a favore della proposta

GIRFATTI *(DCA-PRI-MPA)*. Signor Presidente, signor Ministro, oggi abbiamo ancora una volta l'opportunità di bocciare, come già fatto dalla stessa Commissione europea, l'operato del Governo, di quello regionale regionale della Campania e della intera gestione Bassolino sui rifiuti. Ma a cosa serve oggi bocciare una tragedia annunciata da anni? Infatti si sono sommate, da parte di tutti i commissari, responsabilità gravissime. Omissione ancora più grave, non è stato valutato il disastro ecologico, economico e d'immagine creato ai danni dei cittadini campani e italiani.

Prima di me, lo stesso collega Barbieri, anche nella sua qualità di presidente della Commissione di inchiesta sul ciclo di trattamento dei rifiuti, tra l'altro ha sottolineato le responsabilità degli addetti ai lavori, chiedendo con forza la fine dei commissariamenti stessi. È inutile, quindi, chiedere norme o nuove leggi. Noi rivolgiamo un appello accorato a lei, signor Ministro, e ai rappresentanti del suo Governo

La vostra stagione è finita e i campani sono stanchi. I piani regionali e le proposte serie li avete sempre avuti, ma non avete mai voluto realizzarli ecco i risultati del vostro sistema di potere: in quest'Aula siete stati bocciati da tutti i Gruppi politici e non solo campani. Ancora una volta, risparmiateci le immagini di questi giorni. Tornate a casa, perché siete anche voi campani, anche voi italiani. Non pensate soltanto a sistemare i vostri orticelli e a curare i vostri interessi, come avete fatto per decenni.

valido pensare a questo. Pensate al futuro degli italiani, soprattutto a quello di noi campani, che viviamo oggi in uno stato di assoluta indigenza.

la prova del nove del suo riscatto. Inoltre, siamo consapevoli che il problema della gestione dei rifiuti non è la malattia della Campania ma è un sintomo, seppur il più evidente, ma solo uno dei tanti di una malattia grave e profonda che ne

e di strutture dove si è annidata la malavita; ben venga il passaggio alle istituzioni locali, ma auspichiamo che esso venga attentamente accompagnato dall'unita di crisi e dal Governo perché possa davvero avviarsi quel recupero della dignità morale, ambientale ed etica che tutti ci aspettiamo.

inoltre, ha creato un abisso nel rapporto tra cittadini e istituzioni, non soltanto in Campania

per tutte - la gestione dell'emergenza rifiuti è diventata lo strumento principe di governo, intorno al quale si è creato un vero e proprio sistema di gestione del potere.

il dovere di ricreare un clima di fiducia proprio tra i cittadini e le istituzioni. Per far questo è necessaria chiaramente una svolta. È necessario, come ho già sottolineato nel mio intervento in dibattito generale, rimuovere totalmente e rapidamente tutto il sistema della struttura commissariale.

allo scioglimento dei consorzi, ossia sbaraccare tutta la struttura che in questi anni è cresciuta solo e unicamente su se stessa.

Vorrei soltanto ricordare alcune cifre. La struttura commissariale in questi anni è costata 780 milioni l'anno per consulenze e affitti e solo 29 milioni l'anno per gli investimenti nella gestione dei rifiuti. Detto questo, ricordo al Ministro che è evidente a tutti che per effettuare questa svolta e per chiudere definitivamente con questa impostazione emergenziale (che ha alimentato se stessa, perché l'emergenza creava emergenza), è necessario avere le idee chiare.

Non si può davvero pensare di uscire da questa situazione pensando ancora una volta di trovare delle scorciatoie.

saltando tutti i passaggi che l'Europa ci indica con chiarezza, e che sono gli unici che possono permettere di insediare finalmente un ciclo adeguato di gestione seria ed efficiente dei rifiuti, significa non voler

protrarre le scelte sbagliate che stanno in capo alla situazione odierna. Dobbiamo

Non ci sono gli impianti per una gestione industriale di tutto il sistema della raccolta differenziata. Se si vuole ancora una volta bypassare tutta la questione del riuso, del recupero,

Impregilo. Tra l'altro, ci vorrà tempo per costruire gli altri impianti; non possiamo pensare, in questa situazione di emergenza, in questi centoventi giorni, di non occuparci anche di tutto il resto dell'impiantistica. È incredibile che in tutti questi anni non ci si sia voluti occupare di tali aspetti. Il sistema dell'appalto ha alimentato anche fortemente le penetrazioni camorriste. Vogliamo parlare qui del gioco dei siti

n. 5 a firma dei Capigruppo di maggioranza, ma lanciamo un appello serio al Governo: implementi l'ordinanza per affiancare davvero la possibilità di costruire un ciclo serio ed efficiente per la gestione dei rifiuti, sciolga immediatamente i consorzi, ma soprattutto si arrivi ad una svolta che ridia fiducia ai cittadini e alla popolazione.

da un lato, parlare d'emergenza è del tutto fuori luogo (più che di emergenza, qui si tratta di una telenovela) e, dall'altro, il Governo, anche sul tema dei rifiuti campani, sta dimostrando la sua totale incapacità ad adottare qualsiasi misura.

dei rifiuti, ma ci tengo a ripeterlo sperando che serva a qualcosa. Nel settembre del 2006 i telegiornali di tutto il mondo rilanciano le immagini di Napoli invasa dalla spazzatura. Ormai è diventato un luogo comune: i telegiornali esteri non ne parlano neanche più, perché sanno che questa è la situazione di Napoli e non fa più notizia. Il Governo a notizia. Il Governo a quel punto decide di lanciare in prima linea uno dei suoi uomini migliori: il capo della Protezione civile Guido Bertolaso, il quale praticamente si trasferisce armi e bagagli a Napoli e fa gestire dai suoi uomini più fidati i gangli vitali del commissariato, cominciando a cercare vere soluzioni per il lungo periodo. Fa però un errore: pensa che l'emergenza debba essere risolta, che la telenovela debba finire. Non capisce, Bertolaso, che sulle "scoasse" o sulle "monnezze" (come volete voi) volete voi) di Napoli si è creata un'economia parallela dove la camorra la fa da padrona e, per usare le parole del precedente commissario Corrado Catenacci, festeggia ogni giorno: è dove, praticamente, fioriscono le clientele.

Dapprima Bassolino ne ha a che fare come sindaco di Napoli, come presidente dalla Regione e poi come commissario del Governo, poi solo come governatore. Bassolino non ha perso un solo giorno di emergenza e nel tempo ha permeato il commissariato dei suoi uomini. Bertolaso ha fatto una cosa giusta subito: ha cominciato con il cacciare dal commissariato il vice commissario che risponde al nome di Ciro Turiello, fedelissimo di Bassolino, che è stato però ricompensato con l'incarico di amministratore delegato dell'azienda che gestisce i rifiuti a Napoli.

e ha mandato in prima fila, per gestire il sistema clientelare, il ministro dell'ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio. Bertolaso Bertolaso viene quindi costretto a nominare due vice commissari indicati dal campione dei Verdi: uno risponde al nome di Claudio De Biasio, che viene arrestato negli uffici commissariali per frode aggravata nell'ambito di un'indagine per le infiltrazioni camorristiche del consorzio CE4; l'altro, Alberto Pierobon, viene allontanato quando si scopre che, saputo della sua nomina a vice commissario, aveva costituito una società per la commercializzazione dei rifiuti. Come si vede, quando si tratta di conflitto di interessi ce ne sarebbe da tirar fuori finché si vuole. Fallito il tentativo di ingabbiare Bertolaso con i vice commissari, l'attività di Pecoraro

gran parte dell'emergenza di oggi si deve proprio alla scelta di Pecoraro Scanio, che non ha autorizzato la discarica di Macchia Soprana nella sua interezza. Oggi la Campania avrebbe un sito in cui portare i suoi rifiuti e forse la telenovela avrebbe una certa fine. Ma non è questo che vogliono i Pecoraro Scanio e i Bassolino, che sulla telenovela rifiuti hanno fondato il loro sistema clientelare. Così Bertolaso fa quello che chiunque, con un minimo di dignità, avrebbe fatto al suo posto: se ne va. E al suo posto il Governo nomina il prefetto di Napoli, Alessandro Pansa, il quale punta tutto su un nuovo piano e sull'accelerazione della costruzione dell'inceneritore di Acerra. Il nuovo piano viene presentato,

con tutti coloro che prendono laute prebende per stare nella struttura commissariale, anziché nei loro uffici. Far partire soluzioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti degne di un Paese civile vorrebbe dire lo stop agli stoccaggi e, dunque, la fine dell'assegno mensile che lo Stato è costretto a versare nelle casse degli amici degli amici. Vi anticipo che su questo tema

il prefetto Gianni De Gennaro, affiancato dal generale Giannini. Speriamo che questi uomini si avvalgano anche di esperti della raccolta dei rifiuti e del loro trattamento. Credo infatti

È inutile sperare che l'inceneritore di Acerra sia la panacea di tutti i mali. L'inceneritore, se e quando partirà, risolverà una metà del problema che si risolve solo - è già stato sottolineato da qualcuno, ma bisognerà veramente farlo - con l'avvio di una vera raccolta differenziata, sull'esempio di alcune città del Nord;

Credo che senza immediate risposte a questi due argomenti, purtroppo per noi, purtroppo per il Paese, purtroppo per la Campania e i campani, la telenovela non finirà e continuerà.

il giudizio dell'UDC sulle comunicazioni del Governo è negativo. Non c'è la lucidità d'analisi necessaria per affrontare l'emergenza rifiuti in Campania; è la crisi dei paradossi e dei danni che l'ideologia può provocare se applicata alle tecniche di Governo. In nome dell'ambientalismo è stato prodotto il più grande disastro ambientale nella storia del nostro Paese. In nome della tutela della salute è stato provocato un danno gravissimo alla salute dei cittadini campani, al contrario di quel che ha detto il ministro Turco, smentita da tutta le evidenze epidemiologiche. In nome della lotta alla criminalità è stato consentito alla camorra, che comunque non può essere un alibi, di ingrassarsi con i finanziamenti pubblici ed in nome della tutela e della valorizzazione dell'economia locale sono stati messi in ginocchio il turismo della Regione e le esportazioni dei prodotti agroindustriali. La crisi dei rifiuti è antica, la denunciamo da anni, figlia di una visione arcaica della tecnologia di smaltimento dei rifiuti che la sinistra finto-ambientalista ha utilizzato come strumento d'iniziativa politica. Oggi la Campania è percepita e rappresentata come la pattumiera d'Europa, una sorta di Far West nelle mani di amministratori incapaci e collusi con la criminalità organizzata. Analisti ed osservatori, non a torto, hanno paragonato il disastro rifiuti all'epidemia di colera Il Governo su questo fronte è inadempiente, complice e corresponsabile e, soprattutto, a mio avviso, sottovaluta il problema. Ha bloccato per anni ogni possibile soluzione. L'ostruzionismo scientifico condotto dal Ministro dell'ambiente ha paralizzato la Regione anche quando, come nel caso dell'iniziativa del sindaco di Salerno, è stata chiesta la realizzazione di un termovalorizzatore. Ma la crisi - e questo è il punto, secondo noi - è istituzionale. Il nodo è questo: fino a quando non si capirà la sua vera natura non si potrà avviare a soluzione ed il Governo, purtroppo, in base a quello che ha riferito, non ha coscienza di questa centralità della crisi istituzionale. Il più grande giornale tedesco lo ha detto chiaramente: il problema dei rifiuti in Campania rappresenta una gravissima crisi istituzionale democratica,

Chi si fida più, dopo quindici anni di disastri, delle promesse e degli impegni di Bassolino? Nessuno. Chi può credere ai progetti della Regione per uscire dalla crisi? Nessuno. Se non si sblocca questa paralisi ogni sforzo sarà inutile e né De Gennaro, né San Gennaro potranno fare molto. Per questo occorre partire dalle dimissioni del governatore e del sindaco di Napoli a livello locale e del Ministro dell'ambiente a livello nazionale. Non si tratta di una richiesta propagandistica, né della volontà di colpire i singoli. È solo il tentativo di riattivare partecipazione, fiducia e circuito democratico. Sta qui la soluzione della crisi. crisi. Bisogna ricreare un clima di fiducia e di partecipazione anche tra le forze politiche, per richiamare tutti ai sacrifici che saranno necessari e ancora molto duri. Bisogna ricreare un clima diverso anche nel rapporto tra la Regione Campania e le altre Regioni italiane, così come bisogna

non solo infruttuosa e illogica, ma troppo comoda, così come è comodo e sbagliato - ed è questo il secondo rilievo che muoviamo al Governo e alla maggioranza - minimizzare la portata della crisi che è una crisi di sistema. La Campania è una Regione in coma profondo. L'emergenza rifiuti è solo la punta dell'*iceberg*. La Campania - lo ricordo - è la Regione italiana con il più alto tasso di indebitamento del comparto sanitario (più di 7 miliardi di euro), il più alto tasso di criminalità e, soprattutto, è la Regione europea nella quale un uso sfrenato dei finanziamenti europei non ha portato né a ridurre la disoccupazione, né a far crescere il prodotto interno lordo. È questo il *mix* micidiale che ha portato la Regione allo stremo, al collasso. È una Regione, in sostanza, che lotta per non morire. Noi dobbiamo rianimarla e il Governo mi sembra chiaramente non essere su questa strada giacché indica soluzioni parziali, insufficienti e soprattutto non identifica le vere responsabilità politico-istituzionali che sono alla radice di questa crisi. Non collega le critica alle responsabilità e soprattutto queste ultime ai gesti conseguenti. In questi giorni la stampa internazionale

Siamo arrivati al punto che anche una televisione araba ha potuto rappresentarci come un'area del sottosviluppo e del quarto mondo. Occorre reagire, battere la rassegnazione e non scaricare le tensioni, come purtroppo sta facendo sempre più spesso l'amministrazione della Regione, sulle popolazioni di qualche piccolo paesino paesino delle zone interne, attraverso la "politica delle tre discariche". Come tutti sapete, il gioco delle tre carte è stato applicato allo smaltimento dei rifiuti in Campania, producendo il "gioco delle tre discariche" e questo è davvero inaccettabile. Non mi sembra che questa coscienza Non mi sembra che questa coscienza del problema e di come aggredirlo in termini politico-istituzionali guidi né Bassolino né, tanto meno, il Governo. In Campania il ciclo dei rifiuti non si è mai compiuto.

Signor Presidente, credo che la situazione drammatica che vive la Regione Campania imponga a tutti un senso di responsabilità. Rifondazione Comunista-Sinistra Europea si è assunta il ruolo, in questa fase, di assecondare, in tutti i modi, le scelte del Governo per tentare di risolvere la vergogna dei rifiuti nelle strade della Regione Campania. Questo porta anche ad alcune scelte dolorose, come la riapertura di siti per nuove discariche dopo dieci anni dalla loro chiusura. È chiaramente una scelta grave che va fatta, comunque, nel rispetto della salute dei cittadini e della tutela ambientale. È solo con questa decisione, dolorosa per la Campania, che si può chiedere la solidarietà alle altre Regioni, sapendo comunque che c'è una situazione drammatica rappresentata da oltre 300.000 tonnellate di rifiuti per le strade e che la solidarietà delle altre Regioni darà un piccolo ed importante contributo per poco meno di 100.000 tonnellate. È quindi il momento di avviare seriamente

che tenga conto della gerarchia prevista dalla legislazione comunitaria e internazionale, che interviene su leggi nazionali e regionali, per quanto riguarda la riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata, il riuso e il riciclo e, solo, per la fase terminale, lo smaltimento. Continuare a partire solo con lo smaltimento è un capovolgimento che, come ci dicevano anche i colleghi della Lega, in altre Regioni d'Italia é stato risolto in modo diverso. Ci sono dei punti importanti nelle decisioni del Governo: la fine della gestione commissariale, che chiediamo da anni, e lo scioglimento dei consorzi. Bisogna, però, anche assumere un'altra decisione: occorre interrompere immediatamente la produzione delle ecoballe che hanno

quando dicevamo all'allora ministro Matteoli che quelle ecoballe prodotte non erano a norma e che servivano solamente per alimentare i grandi interessi delle imprese del Nord e dell'Impregilo, non eravamo ascoltati.

veramente strumentale ed immotivata la polemica del presidente della Regione Campania che su un importante quotidiano scrive che la colpa è degli ambientalisti, che hanno bloccato la costruzione dell'inceneritore di Acerra. Di cosa parla? Di cosa parlano gli industriali del Nord? Di cosa parlano i grandi giornali, la destra e anche alcuni interventi che ho sentito in questa Aula da alcuni colleghi del centro-sinistra? La lotta La lotta di Acerra bloccò l'inizio dei lavori per sette mesi. Il 17 agosto del 2004, con l'uso della forza, si aprì quel cantiere, che oggi non si è ancora completato dopo quattro anni e non certo per colpa degli ambientalisti, caro ministro Santagata. Non è colpa degli ambientalisti se quel cantiere non si è portato a termine. Quella lotta, però, portò a galla

degli ambientalisti di quella Regione. Certo, se essi hanno contribuito a dare un impianto più sicuro a quella terra, io rivendico fino in fondo, personalmente e politicamente, la giustezza di quella lotta e di quella battaglia. *(Applausi dal Gruppo* Chi ha lucrato in questi anni in Campania? Dietro la gestione commissariale, che cosa c'era, se non un sistema misto trasversale fra grandi imprese del Nord, settori deviati della politica e dell'amministrazione locale?

di governo di quella Regione. I poteri commissariali hanno invece espropriato gli organi elettivi di qualsiasi possibilità di controllo. Certo, si poteva fare di più e bisogna farlo in queste ore.

bisogna estrometterla anche dagli impianti. Mentre parliamo e i cumuli di immondizia ammorbano la Campania, Impregilo continua ad avere ancora un pezzo importante della gestione degli impianti in quella Regione. non è possibile, dopo l'invio del capo della Protezione civile, del prefetto Pansa e oggi del prefetto De Gennaro. È ora di dire basta! Gli impianti vanno fermati, c'è bisogno di dare un segnale di discontinuità.

della grande impresa, dell'Impregilo, per evitare che questa avesse un tracollo in Borsa. Questo è il vero problema che ha portato a spendere 2 miliardi di euro in quella Regione, per impianti che non sono a norma e un sistema di discariche diffuse su tutto il territorio regionale. Ancora si ripete che gli ambientalisti hanno fermato

sono preoccupato. Sento che nella nuova ordinanza c'è il ritorno di alcuni personaggi che hanno già creato danni in quella Regione. Non vorrei che adesso, con l'atteggiamento - che confermiamo - di collaborazione al prefetto De Gennaro, ci sia un ritorno al passato, si cerchi di violare di nuovo gli accordi che sono stati conclusi con le comunità. Questo sarebbe imperdonabile, metterebbe

In questi anni, si è continuato invece ad assumere decisioni che non andavano in quella direzione, che non affrontavano il nodo strutturale dell'emergenza, ma risolvevano solo il problema visibile dei cumuli di immondizia per strada ed il risultato è quello che abbiamo sotto gli occhi di tutti. Siamo ad sotto gli occhi di tutti. Siamo ad un passaggio importante e c'è bisogno che la città di Napoli dia un suo contributo. Apprezziamo il fatto che nell'ordinanza non ci sia l'indicazione dei nomi delle discariche, ma ci rendiamo conto che la città di Napoli ha bisogno di dare un segnale.

Oltre l'orizzonte dell'emergenza, la Campania segnala però al Paese anche una critica a modelli di consumo e di vita, che sono alla radice di questa crisi di civiltà che attanaglia oggi la Campania e il Mezzogiorno, ma che riguardano

volenti o nolenti, la discussione sull'altra emergenza campana, che anch'essa - come si è visto in questi giorni - è questione nazionale, cioè la crisi della politica campana e soprattutto la necessità di una parola chiara di novità non più rinviabile. Oggi bisogna affrontare l'emergenza non più rinviabile. Oggi bisogna affrontare l'emergenza con il contributo solidale del Paese e gli impegni del Governo nazionale, ma poi bisogna trovare il coraggio per avviare un percorso chiaro di innovazione e partecipazione, prevedendo esplicitamente, prima che lo impongano altri, un deciso cambio di passo. È necessario ridare forza al patto fiduciario tra istituzioni e cittadini nelle forme che sono proprie della democrazia, andando anche oltre le dinamiche dei tempi normali, procedendo con i tempi diversi imposti dalla situazione disastrata che abbiamo di fronte, la quale rinvia ad una vera e propria crisi democratica. É tempo oggi di scelte coraggiose e di chiare assunzioni

oggi di scelte coraggiose e di chiare assunzioni di responsabilità nel dialogo con il popolo campano. Solo così potremo provare ad arginare l'antipolitica e l'offensiva scomposta delle destre, rimettendo sui giusti binari

ma perché avverto il peso del discredito e della vergogna che la vicenda rifiuti ha determinato per la Campania e per l'Italia intera, e perché penso che a volte dovrebbe prevalere il pudore del silenzio e la politica dovrebbe rispondere operando, intervenendo, agendo e concretizzando. Ma poiché c'è ancora una incapacità sostanziale a cogliere la centralità del problema, poiché si fa il richiamo alle responsabilità passate e presenti, con onestà intellettuale di dovere rivendicare una responsabilità e, in particolare, di doverla rivendicare al senatore Matteoli quando è stato Ministro dell'ambiente. Il ministro Matteoli ha una grave responsabilità: quella di avere scritto al Presidente della Regione una nota attraverso la quale contestava l'iniziativa relativa alle discariche e al deposito di ecoballe e nella quale evidenziava l'esigenza che tutto questo fosse a carico dell'impresa FIBE. Quindi, Matteoli ha la responsabilità di avere tutelato l'interesse pubblico nei confronti della speculazione di un privato. *(Applausi ha una responsabilità aggiuntiva: quella di non aver assunto i provvedimenti in via di autotutela suggeriti da quella lettera e da quella nota in nome degli interessi pubblici contro l'interesse di un privato, che ha una chiara responsabilità rispetto a quanto è accaduto, e di un capitalismo straccione che ha le sue responsabilità in quello che è avvenuto in Campania. Ciò detto, mi consentirete però di sottolineare le responsabilità del Governo. Ministro Santagata, ho un sincero apprezzamento nei suoi confronti, ma mi consentirà di sottolineare che la sua relazione è piatta, superficiale ed omissiva. È una relazione omissiva perché salta una scelta del Governo. Capisco la sua difficoltà ad evidenziare un dato che non è ancora emerso in quest'Aula, e cioè che il Governo in carica, prima di nominare il commissario De Gennaro, a dimostrazione di superficialità superficialità e dell'incapacità di cogliere l'importanza del problema, aveva nominato due subcommissari. Siamo passati dal bicommissario al supercommissario. Il Governo aveva nominato il vice prefetto Cimmino e poi abbiamo capito perché: perché: questo funzionario dello Stato doveva assumersi le responsabilità che non si sono assunti il commissario, il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio, e cioè quella di firmare l'ordinanza di riapertura di Pianura. La firma dell'ordinanza di riapertura di Pianura è di Cimmino, a dimostrazione anche di uno stile nell'assunzione delle responsabilità che qualifica, anzi squalifica di per sé il sistema istituzionale, il Governo regionale campano e il Governo nazionale di centro-sinistra. Responsabilità. Carissimo signor Ministro,

ha stigmatizzato le scelte del Governo dal punto di vista normativo, ad iniziare dal decreto-legge poi convertito in legge, ritenendole inefficaci rispetto al problema.

nell'attività di smaltimento dei rifiuti non deve, secondo il Commissario, rappresentare per il Governo italiano un alibi rispetto all'attuale situazione di emergenza, la cui diretta causa essere l'inerzia e la mancanza di volontà politica nell'adottare le misure necessarie a risolvere il problema della gestione dei rifiuti.". Il problema dei rifiuti in Campania

maggioranza il dibattito parlamentare in sede di conversione del decreto-legge. La prima relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti situava al mese di ottobre la data in cui realizzare l'accordo di programma quadro e l'intesa istituzionale per determinare la filiera della responsabilità in Campania, chiamando dunque il Governo nazionale, la Regione, le Province e i Comuni capoluogo ad assumere impegni chiari e definiti nell'individuazione dei siti, nella percentuale di raccolta differenziata, nella tecnologia e nell'impiantistica necessarie per il ciclo industriale dei rifiuti. Noi chiediamo autonomia e responsabilità.

«non chiedere mai agli altri quello che non hai prima chiesto a te stesso». In Campania bisogna prima chiedere a noi stessi lo sforzo di responsabilità e di autogoverno e poi chiedere la solidarietà nazionale. *(Applausi un'intesa istituzionale di programma e poi chiedere alla Conferenza Stato-Regioni di sottoscriverla perché i campani si impegnino a scegliere i siti per le discariche per tre anni, a completare l'impiantistica dei termovalorizzatori e a determinare una percentuale di raccolta differenziata.

Signor Presidente, qui è in discussione un modello, la pretesa del centro-sinistra di avere un modello egemonico in Campania come sul piano nazionale. Nella musica e nella cultura, mettendo insieme Pino Daniele e i neomelodici, nel teatro, mettendo insieme Martone e Rivieccio, mettendo insieme tutto e il contrario di tutto e mettendo insieme l'alleanza che passava come anticipatrice sul piano nazionale dei centri sociali e del centro mobile, di Caruso e di Mastella, tutto tranne la capacità di governare. Questo è il tema, questo è il problema, questo è il fallimento.

Stiamo assistendo ad un dibattito articolato e delicato che coinvolge, secondo noi, responsabilità di questo Governo. Lo abbiamo chiesto: mercoledì discuteremo la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Pecoraro Scanio. Questo dibattito si è dilungato al di là degli orari previsti, dei quali tutti i parlamentari erano a conoscenza.

ma perché dobbiamo darci un obiettivo: quello di essere un palazzo di vetro e trasparente. Se avalliamo una ipotesi di sforamento

Riteniamo che la Presidenza, nella logica delle regole fondamentali del nostro funzionamento, debba sospendere la seduta - se lo riterrà e noi lo chiediamo lo chiediamo - per una questione di trasparenza e non perché non vi sia la volontà di votare che, anzi, abbiamo chiesto noi. Tra l'altro, credo che questo dibattito si stia svolgendo in piena serenità, seppure nella conflittualità dello scontro politico. Ma le regole sono regole. Siamo disponibilissimi a continuare questo dibattito nella giornata in cui deciderà la Presidenza, anche all'apertura della seduta di martedì prossimo, per continuare a discutere di questo tema con eventuali integrazioni ed interventi, facendo in modo che tutto avvenga nel rispetto della compostezza e dei paradigmi che ci siamo sempre dati,

non altro. Non credo che dobbiamo attaccarci ai pochi minuti che mancano. Per il rispetto delle regole i senatori sapevano che si sarebbe votato stamattina. Quindi, si sono adeguati e regolati in questi termini. Non credo che vi siano senatori in Aula in questo momento con l'orologio in mano per prendere l'aereo delle ore 14 piuttosto che quello delle 15. Il nostro primo dovere è quello di stare in Aula a votare. Questa è la decisione presa all'unanimità nella Conferenza dei Capigruppo.

Noi abbiamo delle regole, che fissiamo in Conferenza dei Capigruppo. Ove votassimo questa proroga, lei creerebbe un precedente, quello di consentire ad una maggioranza d'Aula, all'ultimo minuto (tra l'altro alla scadenza della seduta, perché questa in teoria è già terminata e la proroga andava chiesta in mettere in votazione la proroga di una seduta di Aula appunto già scaduta. Se si votasse una cosa del genere si consentirebbe per il futuro a qualunque maggioranza, e dico qualunque maggioranza, di fare quello che vuole sulla durata delle sedute parlamentari.

perché, in teoria, l'Aula è sovrana. Attenzione, signor Presidente, perché la logica dell'alternanza ci pone ad essere oggi opposizione e domani maggioranza e ad essere trasversali nel modo di pensare.

e che si avvalgono del principio dell'affidamento dei terzi, ritengo che un mutamento di queste regole soltanto con un voto dell'Assemblea creerebbe un *vulnus* per il futuro che noi vorremmo evitare. Ribadiamo che siamo prontissimi a votare, non abbiamo nessun problema, perché si tratta di un tema che riguarda squisitamente la trasparenza e le regole, quelle che

Presidente, la discussione che abbiamo svolto, che tra l'altro ha evidenziato posizioni diverse all'interno della stessa maggioranza, ha configurato un dibattito importante e ricco per le conseguenze che la questione dei rifiuti in Campania può avere anche per il futuro della gestione stessa dei rifiuti.

Presidente, prima di tutto voglio chiedere al collega Ripamonti come si fa a parlare di divergenze nell'opposizione se qualcuno chiede

Presidente, capisco che lei possa decidere o meno se votare ora e mi rimetto al suo buonsenso; comprendo anche coloro che sono intervenuti dicendo che è opportuno votare, poiché si è sforato di poco. L'unica cosa inaccettabile è che lei metta ai voti la possibilità di continuare o meno, perché ciò è assolutamente inaccettabile. mi rimetto a lei: se deciderà di votare, il Gruppo di Alleanza Nazionale sarà qui a votare, altrimenti non avremmo più la certezza dei lavori nell'Aula del Senato e questo non lo possiamo assolutamente accettare.

ma soprattutto non scritte, nel comportamento tra di noi, nella vita interna di questa Camera di eccellenza del nostro Paese. Se non rispettiamo nemmeno queste norme minime di convivenza e di *bon ton* nel Senato della Repubblica credo che, signor Presidente, apriremmo un precedente veramente disdicevole. Pertanto, per

Lei si sta assumendo la responsabilità di far votare l'Aula al di là dell'orario prefigurato? Questo le sto chiedendo.

Bene, Presidente, noi ci riserviamo ogni atteggiamento in occasione del voto, perché non ci risulta che sia successo in passato che la Presidenza abbia assunto una decisione con un'Aula divisa su un tema così delicato.

di comica gestualità decisionale? Perché è comico un Presidente del Consiglio che con decisionismo sudamericano dalle televisioni di Stato ed anche private annuncia che nell'arco di ventiquattro ore l'Esercito riaprirà le scuole. Forse credeva di essere il generale Videla in Argentina.

affermato che i soldati si sostituiranno agli spazzini per ripulire Napoli e che comunque la discarica di Pianura sarebbe stata riaperta. Naturalmente, nessuno di questi annunci è stato seguito da fatti concreti. In realtà, si tratta soltanto di gride manzoniane, ma siccome in quest'Aula da anni si mente sulle origini di questa emergenza rifiuti, è giusto fare il punto su che cosa sia avvenuto fin dal 1994. Presidente, nel 1994 la Campania era governata da una Giunta di centro‑sinistra sostenuta dall'allora Partito Democratico della Sinistra che vantava anche presenze determinanti, come il controllo dell'assessorato alla sanità.

chiese a Rastrelli di seguire un'altra strada, quella del bando europeo. Rastrelli accetta il suggerimento ed ecco che sette società partecipano alla gara. Perché vince l'Impregilo? Nel bando di gara si prevedeva anche la capacità di un polmone finanziario per costruire questi termovalorizzatori che altre società non avevano.

mette in crisi la giunta Rastrelli e nel 1998 l'allora presidente Losco dell'UDC,

Successivamente, è il presidente Bassolino - ma voi queste cose non le dite - a firmare materialmente l'accordo con l'Impregilo; non è Rastrelli e nemmeno Losco, è Bassolino che firma l'accordo con l'Impregilo. Perché Bassolino poi permette all'Impregilo di fare il buono e il cattivo tempo? Per un motivo semplicissimo: perché Impregilo significa famiglia Romiti, Romiti, dunque il sostegno de "La Stampa" e del "Corriere della sera", oltre al sostegno pregiudiziale de "la Repubblica"; quindi significa anche il sostegno di

Queste sono responsabilità che dovevano portare non solo gli assessori alla sanità e all'ambiente, ma anche il Presidente della Giunta in galera se a Napoli ci fossero stati dei magistrati degni di questo nome.

i magistrati, dopo una sospensione del CDR di Santa Maria Capua Vetere di qualche giorno, si guardarono bene dall'aprire un'inchiesta, e non a caso. Sapete, infatti, chi era il magistrato competente per i reati in materia ecologica?

dove lavora ora il magistrato che ha scoperto questo scandalo? È stato costretto ad andare via, ad abbandonare la distrettuale la distrettuale antimafia ed ora siede in Cassazione. Sapete cosa accade a Napoli, quando il procuratore Cordova solleva la pietra che nasconde il verminaio della gestione emergenza? Avviene che

che governavano ed anche con i magistrati collusi con i sistemi criminali, come il capo di questa insubordinazione in procura della Repubblica, che era

Presidente).* Questo è il quadro. Questo è il contesto politico‑criminale. È un magistrato che osa dire: guardate che Mancuso frequenta abitualmente criminali e fiancheggia...

Mi sto richiamando ad una denuncia del magistrato Corona che è stata insabbiata dalla procura di Roma. Sto parlando di un *kombinat*, di un contesto

L'eventuale approvazione della proposta di risoluzione n. 1 determina effetti di assorbimento nei confronti delle proposte di risoluzione nn. 6 e 7 nelle parti relative allo scioglimento del Consiglio regionale della Campania. Viceversa, la reiezione del medesimo strumento precluderà le proposte di risoluzione nn. 6 e 7 per le parti di analogo contenuto relative al Consiglio regionale della Campania.

Ciò in quanto le proposte nn. 3 e 4, pur menzionando la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, fanno riferimento ad aspetti non confliggenti e comunque tra di loro compatibili. di risoluzione nn. 3 e 4 hanno contenuti del tutto analoghi tra di loro, salvo il riferimento contenuto nella premessa del secondo di tali testi alle responsabilità delle amministrazioni regionali. Pertanto, dopo la votazione della proposta di risoluzione n. 3 verrà posta ai voti anche la successiva n. 4 nelle parti non assorbite. La proposta di risoluzione n. 5, dopo avere nella premessa sostanzialmente ripetuto contenuti largamente condivisi dai testi precedenti, nella parte dispositiva approva il contenuto delle comunicazioni del Governo. Verrà pertanto posta ai voti, qualsiasi sia l'esito delle votazioni precedenti. In caso di approvazione della proposta di risoluzione n. 5 risultano precluse le proposte di risoluzione nn. 6 e 7 nella parte relativa alle responsabilità del Governo centrale contenuta nelle premesse. Verranno quindi poste ai voti nelle restanti parti. Resta salvo quanto già comunicato circa gli effetti di preclusione ed assorbimento relativi alla proposta di risoluzione n. 1.

al punto che lei stesso ha dichiarato che l'eventuale reiezione determinerebbe una preclusione. Proprio per superare anche questo aspetto, e quindi non rendere preclusi

Signor Presidente, con riferimento all'indicazione venuta dal senatore Calderoli e tenendo presente che la premessa della sua proposta di risoluzione parla di «estrema pericolosità e gravità per la sicurezza nazionale», considerato che il terzo passaggio dell'impegno fa riferimento all'articolo 126 della Costituzione, che prevede proprio il tema della sicurezza nazionale come una delle tre fattispecie per le quali si può proporre la rimozione del Presidente della Giunta, a me pare che, al fine di evitare ogni possibilità di equivoco tra il riferimento all'estrema pericolosità e gravità per la sicurezza nazionale, che è in premessa,

Senato non approva.**

colleghi, comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri renderà una informativa urgente sulle dimissioni del ministro della giustizia

nel riferirsi ad una mia lettera, la lettera di dimissioni di cui avremo modo di parlare ritengo tra breve in quest'Aula, possedendo evidentemente doti divinatorie - quella lettera nella sua interezza non è mai stata resa pubblica - ha confuso il medico con la malattia e mi ha confermato tra parentesi

scrivo che le mie dimissioni sono motivate proprio per difendere le istituzioni dalla deriva di sfiducia che investe la politica. È evidente poi, Presidente (basta leggere i giornali di oggi), che la semplificazione mediatica che viene fatta complessivamente di un ceto politico che, di fronte a ciò che è avvenuto in questi ultimi tempi e ieri in particolare, si arrocca in una difesa sterile della sua autorappresentazione, non può che essere quella, come oggi titolano diversi giornali, della casta. Non è certo colpa di chi indica il male